finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

È stato ovviamente un piacere poter lavorare con colleghi che sono stati sindaci di alcuni Comuni colpiti dal terremoto

e anche alcune parti fiscali più pesanti che hanno necessità di fondi veramente ingenti, non sono state bocciate dal Governo perché non interessano o perché non sono considerate

questi due, in particolare, attualmente sono ancora aperti e su di essi ci stiamo veramente mettendo attenzione, perché richiesti a larga maggioranza.

gli emendamenti 1.65, 1.0.103, 1.0.104, 1.0.120, 1.0.122, 1.0.127 e 1.0.128, in quanto recano disposizioni estranee

G1.2, relativo alle aree che attualmente ospitano le strutture abitative di emergenza, che sono utilizzate in forza di contratto di locazione. Ebbene, con questo ordine del giorno chiediamo al Governo di valutare la possibilità che, nell'ambito di un prossimo provvedimento, si possano stabilire le acquisizioni, attraverso l'esproprio, delle aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza, nonché

su tante aree presenti in molti Comuni del cratere che necessitano di una programmazione. Illustro, poi, gli analoghi ordini del giorno G1.300 e G1.301, che riguardano la rateizzazione della busta paga pesante. L'attuale decreto-legge la proroga del termine oltre il quale bisogna restituire i versamenti tributari e i contributi assicurativi previdenziali al gennaio 2019 e pone in 60 rate la restituzione

dei versamenti tributari a 120 rate - e questo è previsto nell'ordine del giorno G1.300

Ebbene, noi riteniamo che, al fine di alleggerire il peso della doppia tassazione cui andrebbero incontro i cittadini privati, sarebbe opportuno pensare, nella prossima legge di bilancio, a una rateizzazione

l'assunzione a tempo determinato del personale oggi impegnato presso i quattro uffici speciali della ricostruzione, associati alle quattro Regioni colpite dal terremoto, e

dai Comuni: i Comuni del cratere sono sempre più spesso impegnati nel dover affrontare una serie di spese legali che scaturiscono da procedimenti amministrativi o penali derivanti dalla gestione dell'emergenza

o di strutture pubbliche di servizio, di procedimenti di verifica e revoca del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS), dell'assegnazione e della revoca del contributo

adottare iniziative per la creazione di un fondo specifico per i Comuni del cratere destinato al sostegno delle spese legali - sono tante e saranno sempre maggiori - per fronteggiare siffatti contenziosi.

G1.312, che riguardano sostanzialmente la zona franca urbana, ha stabilito il diritto a una serie di esenzioni da parte delle imprese. Il problema è che dette esenzioni, che non sto qui ad elencare, sono stabilite in base a una diminuzione del fatturato che le imprese hanno registrato nell'ultimo periodo del 2016

ha diritto a una serie di esenzioni. Peccato che molte imprese colpite pesantemente dal terremoto, anche grazie alla solidarietà

tenuto un fatturato alto, che poi nei primi mesi del 2017 è andato scemando. Con questi due ordini del giorno chiediamo al Governo di rivedere

trattabile - e di rivedere l'arco temporale oggetto di confronto dei fatturati delle imprese che hanno avuto nocumento dal territorio.

Un provvedimento preparato dal Governo Gentiloni Silveri, che lo ha licenziato come suo atto, e in questo c'è

ai sindaci e ai soggetti sociali ed economici del cratere, ma dell'importanza politica che si è voluto dare a questo tema. esame è un decreto-legge che, nonostante la preparazione ampia, alla fine è rimasto circoscritto nel testo approvato in Consiglio dei ministri il 29 maggio, in prossimità della scadenza della sospensione dei tributi - dei tributi - alla proroga dei termini relativi ai tributi e ai versamenti contributivi, alla proroga di uno strumento fondamentale che abbiamo voluto per proteggere il reddito e sostenere le esigenze economiche dei lavoratori,

presto e bene, i muri, le case; la vinceremo soprattutto dando un progetto a quei territori colpiti anche da una lunga crisi economica, e quindi deboli. Progetto significa innanzi tutto lavoro, sostenere le imprese, sostenere i distretti industriali del manifatturiero, dell'agroalimentare, dell'artigianato che in quei territori insistono e che sono tra le eccellenze italiane. La gran parte dei nostri emendamenti, colleghi, riguarda questo: la semplificazione amministrativa, il sostegno alle imprese, anche quelle piccole, anche quelle artigiane; prorogare una mole di provvedimenti che in dichiarazione di voto presenteremo uno ad uno; aiutare i sindaci, soprattutto quelli dei piccoli Comuni, a trovare personale per

bocciata dalla maggioranza e dal Governo, e questo è un rammarico enorme che rischia di vanificare le attese. Non è un no agli emendamenti del PD; è un no alle istanze dei territori. Ripresenteremo quegli emendamenti e li illustreremo uno ad uno, con l'auspicio che quest'Assemblea davvero possa farli propri, perché altrimenti, in un momento cruciale della ricostruzione post-sisma,

che in questi due anni, tra mille difficoltà, il Governo Renzi, prima, il Governo Gentiloni Silveri, poi, i sindaci, le Regioni, tutti i parlamentari - sono atti sui quali tutti abbiamo lavorato insieme - hanno contribuito a fare. Non vogliamo tornare indietro, presenteremo i nostri emendamenti facendo un appello fortissimo al Governo e alla maggioranza perché li accolgano per il bene dei territori e delle popolazioni che attendono risposte.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non vorrei disilludere il collega del PD che poc'anzi ci richiamava alla

alla proroga delle agevolazioni fiscali per i residenti nell'area del cratere. È stata scelta dal nuovo Governo la formula formula opinabile, ma comunque dal mio punto di vista condivisibile, di approfittare dell'occasione per affrontare l'enorme massa di problemi che ci trascinavamo dietro dalle vicende dell'emergenza ad oggi, determinate evidentemente dalla parziale azione del precedente Governo (nel dire parziale sono molto buono). Questa è stata, all'inizio, un'operazione che noi abbiamo condiviso. Insieme al collega Marsilio abbiamo partecipato attivamente ai lavori della Commissione e devo riconoscere che essa ha affrontato con lo spirito giusto tutte le tematiche riguardanti la ricostruzione e, provenendo dal territorio del cratere, posso affermare che gran parte delle problematiche emerse in questi due anni sono state evidenziate, affrontate e, in qualche caso,

Abbiamo parzialmente affrontato soltanto le operazioni che non prevedevano spesa, sono state cassate proposte ritenendole prive di copertura e abbiamo dovuto aspettare le relazioni tecniche per capire di quali coperture si parlasse. Nella sostanza, Fratelli d'Italia intende riproporre in Aula

l'elemento più interessante di questi giorni di lavoro sul decreto terremoto, cioè lo spirito con cui il Senato ha ritenuto di affrontare queste problematiche. Spero che ciò si traduca, Presidente, in

d'intesa tra il commissario straordinario, la Protezione civile e il Comune. La vicenda, purtroppo, ha visto l'invio di avvisi di garanzie e l'iniziale sequestro della struttura. Chiediamo al Governo di valutare l'applicazione di quanto previsto dall'ordinanza anche per le strutture

parere favorevole

parere contrario,

per svolgere una dichiarazione di voto complessiva, onde evitare di intervenire su tutti gli emendamenti. Apprezzando il lavoro che tutti insieme abbiamo svolto in Commissione, voteremo gli emendamenti approvati in quella sede, compreso l'ultimo presentato dal relatore. Non voteremo tutti gli altri emendamenti per una ragione semplice: non perché non condividiamo tanti di quegli emendamenti, ma in virtù del lavoro svolto dalla Commissione e dell'impegno assunto dal Governo di affrontare una serie di altri provvedimenti nella legge di bilancio.

importante, quello della tutela dei diritti delle persone diversamente abili, prevedendo, quindi, oltre all'adeguamento igienico, sanitario, energetico e antincendio, anche l'eliminazione delle barriere architettoniche. Non occorre, quindi, che mi dilunghi oltre, se non per ricordare che le sofferenze patite dai cittadini colpiti dal sisma

parere contrario

parere contrario

*(FdI)*. Questo emendamento riguarda una materia già trattata peraltro dal collega Arrigoni, con la trasformazione del suo emendamento in un ordine del giorno.

Anche questa è una norma di civiltà, oserei dire. Nel momento in cui vengono riconosciute delle agevolazioni in virtù di uno stato di emergenza, quelle agevolazioni non possono essere rimborsate finché permane lo stato d'emergenza stesso. Capisco anche qui le difficoltà di provvedere a una sistemazione tecnica della copertura,

Ieri abbiamo ascoltato diversi interventi da parte di altre forze di opposizione e della maggioranza, che sostanzialmente condividevano lo spirito di questo emendamento. Del resto, è stato fatto un prezioso lavoro in Commissione speciale, che proseguiva quello significativo e importante svolto dal precedente Governo, in una fase peraltro complicata e difficile; Governo che pure è stato in grado di approntare un provvedimento che finalmente potesse dare ulteriori risposte alle terre colpite

di queste comunità. I sindaci di queste terre sono venuti in Commissione e hanno posto con forza la necessità di intervenire. Noi, come Partito Democratico, abbiamo fatto nostra la loro voce, che chiede

giunti al momento in cui passare dalla propaganda alle risposte concrete. Il Partito Democratico vi chiede di lasciare il terreno della propaganda e di fornire risposte concrete, guardando alle esigenze di queste comunità. Ve lo chiediamo facendo appello al senso di responsabilità. Non comprendiamo il passo indietro che qualcuno è disposto a fare, di fronte alla richiesta del Governo

sicuramente minerebbe la ripresa in maniera considerevole. Vi chiediamo di non sprecare questa importante opportunità che possiamo costruire insieme. Vi chiediamo di non venire meno a impegni che avete assunto anche voi. Vi chiediamo soprattutto di sostenere in questo caso l'appello del Partito Democratico a votarli e a farlo adesso. Nessun rinvio, che non si comprenderebbe, e nessun rinvio sulla pelle dei territori del Mezzogiorno, e in questo caso di un'isola come Ischia,

Anche noi, come Gruppo Forza Italia, abbiamo lavorato in sinergia per avviare il percorso della ricostruzione, come ho già detto ieri nel mio intervento, al fine di creare le condizioni concrete affinché ciò possa essere reale, con la nomina del commissario e quant'altro. Il Governo e i partiti che sostengono questa maggioranza hanno ritenuto di prendersi un lasso di tempo per poter meglio elaborare e valutare le proposte che sono venute da Forza Italia e dal Partito Democratico. Essi hanno assunto l'impegno,

poi, alla collega del Partito Democratico che il terremoto di Ischia si è verificato il 21 agosto 2017 e che, dopo quella data,

il Governo Gentiloni Silveri, senza dare risposte alle comunità di Ischia, è intervenuto con il decreto fiscale di ottobre e con la legge di bilancio 2018 del dicembre dello scorso anno. *(Commenti della su Ischia, d'accordo con tutti i Gruppi della Commissione speciale, abbiamo ritirato gli emendamenti per convergere su un ordine del giorno.

finalmente si parla anche dei piccoli Comuni dell'isola d'Ischia, che nell'agosto 2017 hanno subìto un evento tragico. Il disegno di legge

all'interno una normativa a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

delle norme e degli impegni per Ischia. Abbiamo fatto sì che i sindaci di quel territorio venissero finalmente in Senato a parlare dei loro problemi

Ma sappiamo benissimo - e lo sanno tutti i colleghi di quest'Assemblea - che questo decreto-legge, scritto dal Governo Gentiloni

perché c'è un difetto di copertura secondo la Commissione bilancio. Il Parlamento può votarlo comunque, anche in presenza di tale difetto, ma ferme restando

Signor Presidente, questo emendamento ha grande rilevanza, perché si occupa del sostegno economico alle imprese. Governi del Partito Democratico, come mai prima era avvenuto per un sisma, hanno riservato al tema del sostegno economico alle imprese una grandissima rilevanza. Abbiamo introdotto una misura molto forte, molto utilizzata, che ha

chi vota contro questo emendamento vota contro la prosecuzione dell'*una tantum*; vota oggi contro le imprese che ne hanno bisogno. È oggi che si fanno le scelte: chi poco fa ha votato contro Ischia ha votato contro Ischia; chi poco fa ha votato contro l'emendamento che anche noi proponevamo per allungare le rate dei mutui e dei pagamenti sospesi da 60 a 120, appena votato contro un aiuto alle popolazioni del terremoto. Allo stesso modo, quando voteremo per decurtare l'importo da restituire - come noi abbiamo proposto - fino al 40 per cento, chi voterà contro farà oggi una scelta contro il sostegno alle popolazioni del terremoto. Signor Presidente, le scelte si fanno oggi in quest'Assemblea. Il decreto-legge licenziato dal Consiglio Ministri era circoscritto, perché il Governo era dimissionario - e solo per quello - ma abbiamo assunto l'impegno tutti insieme di ampliarlo, a partire dallo sforzo che abbiamo fatto con il commissario De Micheli. Assumetevi le vostre responsabilità: non fuggite e votate oggi a favore o contro le imprese, a favore o contro questo emendamento.

Presidente, colleghi, fino ad oggi più di 1.500 giovani hanno avuto la possibilità di fare un'esperienza di volontariato, rinsaldando il vincolo di solidarietà e aiutando popolazioni in grande difficoltà.

per i territori, per le popolazioni colpite e soprattutto resterà per questi giovani che matureranno la loro coscienza di cittadini nel modo più alto, aiutando chi, con il terremoto, ha perso tutto. Chiediamo quindi che questo emendamento venga votato e approvato. *(Applausi dal Gruppo

uno dei temi è quello del personale per i Comuni, per rispondere alle esigenze *post* sisma. Uno dei temi è anche quello di concedere ai Comuni la possibilità di assumere agenti di polizia locale

Quello che abbiamo sostenuto in Commissione e che poco fa ricordava il collega Verducci è relativo ai Comuni, quindi al territorio e alle amministrazioni locali che esattamente dal 1° di agosto, perderanno

La stessa cosa vale per gli agenti di polizia municipale e per le deroghe fin qui ottenute. Quindi l'obiettivo era quello. L'ho detto in Commissione e sono sicuro che nessuno sia contrario a questo punto di vista, però secondo noi era necessario fare uno sforzo, peraltro modesto dal punto di vista finanziario, che avrebbe consentito ai municipi, alle amministrazioni locali ed ai territori di poter continuare il lavoro fin qui portato avanti. Dal 1° agosto tutto ciò cesserà, quindi noi voteremo a favore dell'emendamento 1.56 e ovviamente anche del nostro che successivamente sarà posto in votazione. ovviamente legata allo stato di emergenza che verrà prorogata ulteriormente con un dispositivo che il Governo prenderà in considerazione anche nella legge di bilancio, quindi questa situazione verrà prorogata anche nel 2019. Per quanto riguarda, invece, il personale degli UTR, cui forse faceva riferimento il collega, la scadenza è il primo luglio, non

di rafforzare la capacità degli enti locali di dare risposte alle tante esigenze di istruttoria amministrativa e tecnica in questa importante fase della ricostruzione.

(visto che il terremoto aveva colpito quattro Regioni e, quindi, si ravvisava questa necessità), affiancato da quattro vice commissari, presidenti di Regione, e dagli uffici speciali. In questa ulteriore fase fase - attuativa - della ricostruzione è necessario rafforzare gli enti più vicini ai cittadini, cioè i Comuni, affinché trovino risposta le diverse esigenze che riguardano la parte privata, la ricostruzione edilizia, ma anche le richieste delle imprese per quanto riguarda le delocalizzazioni e

ricrea il senso di comunità del territorio. È necessario rafforzare questa capacità di dare risposte, così da ridare fiducia a quelle popolazioni che hanno scelto di continuare a vivere in questi territori. Stiamo parlando di popolazioni estremamente laboriose, che hanno dimostrato una grande

il Governo sia in grado di dare queste risposte, su cui noi richiamiamo l'attenzione.

questo emendamento, che è teso a prorogare la zona franca urbana, che prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. È un atto fondamentale per sostenere la ripresa economica delle zone colpite dal sisma. L'introduzione della zona franca urbana - lo sanno bene tutti i colleghi del territorio delle quattro Regioni colpite - è una vittoria che abbiamo conseguito nei mesi precedenti dopo

dell'Aquila del 2009 e del proseguimento delle normative per il sisma 2012 che invece ha colpito la Regione Emilia. Con l'emendamento 1.86 di cui avrei dovuto parlare, coerentemente e Grazie,

Presidente, la gran parte dei Comuni del nostro cratere è fatta di Comuni molto piccoli, di zone montane e di zone collinari. Comuni piccoli che molto spesso hanno difficoltà, per il contesto particolarmente difficile, ad avere dei segretari comunali. La figura del segretario comunale è decisiva per rispondere alle esigenze del terremoto. Noi chiediamo di riclassificare le sedi di segreteria comunale per i municipi del cratere

è in difficoltà: c'è un piano industriale minaccioso, con addirittura il rischio di 131 esuberi e che andrà respinto a partire dal 6 luglio, quando ci sarà la prima riunione al Ministero dello sviluppo economico. C'è però un primo tema, quello degli ammortizzatori sociali, che stanno con questo emendamento il Partito Democratico ha voluto portare in Parlamento la questione della Whirlpool. Abbiamo chiesto le certezza per gli ammortizzatori sociali per ventiquattro mesi; la prima vittoria a sostegno dei lavoratori per una vertenza più complessiva. Ci è stata accordata per soli sei per soli sei mesi, ma è comunque una prima vittoria che ci consentirà di legare a questa vertenza quella per un progetto per il territorio. È un emendamento che ci inorgoglisce,

con questa battaglia, colleghi, sperando di trovarvi tutti in un fronte unitario a sostegno di questa azienda, a sostegno del lavoro e a sostegno dei Comuni e del territorio colpiti. *(Applausi

è un lavoro che è stato già fatto a favore dei Comuni e che tutto ciò per cui si è trovato uno stanziamento, al fine di dare sollievo a questi Comuni, lo si è già fatto.

nel frattempo le amministrazioni comunali hanno una difficoltà enorme, perché piccoli Comuni si ritrovano a fare un lavoro enorme, sproporzionato alle loro competenze tecniche e alla struttura amministrativa di cui possono godere.

dedicate al servizio di quei territori, perché o si potenziano queste strutture oppure non si sblocca la ricostruzione, in quanto semplicemente i pareri restano fermi, non si concludono le procedure, non si va a gara sempre per questa ragione. Quindi pensiamo la struttura dell'ANAC e decentrarla sul territorio, in una condizione di straordinarietà e di emergenza, come quella che caratterizza la vicenda del terremoto, del terremoto, sia una misura necessaria e utile per aiutare le amministrazioni a fare meglio, più velocemente e più tempestivamente il loro lavoro.

intervengo per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.122, condividendo pienamente le motivazioni ora esposte dal senatore Marsilio e invitando il Governo, nonché il relatore, a riflettere in termini generali

e ci mancherebbe), tuttavia ci sono degli aspetti procedurali che vengono sottovalutati e questo è uno di tali aspetti fondamentali. ha introdotto delle procedure e di questo discuteremo un'altra volta; c'è stato un accenno di discussione anche da parte del nuovo Governo, che è poi subito rientrato non appena Cantone si è espresso. Per carità, nessuno critica l'ANAC perché tifa per la corruzione, ma perché c'è un problema di funzionalità dei controlli e degli interventi;

per far funzionare le iniziative di ricostruzione. Pertanto, ho colto l'occasione di questo emendamento non solo per dichiararmi a favore, ma anche per invitare a riflettere sull'altra questione inerente al personale, che è stata prima affrontata con motivazioni infondate infondate ed errate. Mi hanno impressionato più le motivazioni che il diniego, perché non si percepisce quello che accadrà. Tutti vanno poi a farsi i *selfie* coi sindaci: facciamo gli emendamenti per i sindaci, non i *selfie.*

degli ordini del giorno G1.3, G1.4, G1.301, G1.5, G1.316, G1.8, G1.309

assolutamente banale e, cioè, al calcolo della superficie utile per l'ottenimento del contributo per la ricostruzione. Vi sono differenze edificative sostanziali tra territori diversi. Faccio solo l'esempio del prevalente utilizzo di materiale laterizio nell'Emilia, e in parte nel Lazio, e del prevalente utilizzo della pietra a secco in Umbria e nelle Marche. Questa vicenda induce a dover ritenere la superficie utile per il calcolo del contributo quella perimetrale esterna,

per quale motivo si dovrebbe mantenere tale disparità di trattamento.

Grazie,

è frutto di un lavoro comune svolto in Commissione. Il senatore Arrigoni, che mi osserva, ha presentato un testo Grazie,

si tratta delle modalità di ricostruzione degli edifici di culto, delle chiese, nelle aree terremotate. Come potete immaginare, al di là di basiliche e di chiese che sono importanti monumenti - pensiamo a San Benedetto a Norcia - che hanno suscitato l'attenzione internazionale e spesso anche interventi di organismi come l'Unione europea (il Presidente del Parlamento europeo Tajani annunciò iniziative proprio relativamente alla celebre chiesa di San Benedetto a Norcia), ci sono migliaia di chiese sparse sul territorio che sono punto di incontro, di ritrovo delle comunità e, al di là del pregio artistico maggiore o minore che possono avere, sono importanti. Noi avevamo posto la questione, che è stata oggetto anche di un'audizione in Commissione speciale dei rappresentanti della CEI. La richiesta verteva sulle procedure nel senso che se gli edifici di culto vengono considerati edifici pubblici, tutte le procedure e gare di appalto rendono impossibile o lentissima la ricostruzione. Certamente bisogna dare ai cittadini una casa ma anche una chiesa in una comunità, soprattutto le più sparse e sperdute, è un punto di incontro, di aggregazione e di socialità, oltre che per chi, come il sottoscritto, è credente, anche un valore spirituale. Questo emendamento frutto della Commissione consente, al di sotto di una certa soglia - 500.000 euro - di garantire procedure simili a quelle di una ricostruzione privata, come se fosse la ricostruzione di una casa per la quale il privato, ovviamente, avrà i contributi, se ne avrà diritto, ma potrà seguire procedure semplificate senza dover fare gare d'appalto come se fosse la prefettura, la questura o altri edifici che ovviamente seguono altre logiche. Questo emendamento, quindi, è frutto del confronto, delle iniziative che il nostro Gruppo aveva

Faccio intanto curiosamente notare che l'Assemblea, con il voto dei 5 Stelle, ha appena respinto l'emendamento che puntava a istituire il reddito di cratere per la gente che vive in quei territori che non ha più un lavoro perché non esiste più l'attività con la quale potevano vivere mentre qualcuno pensa di dare un reddito di cittadinanza a chiunque e dovunque, noi, che riteniamo sbagliata quella misura, la ritenevamo invece utile per chi oggettivamente è nella condizione di non poter lavorare. Va bene, questo lo abbiamo visto. Ora, l'emendamento 1.0.24 di adoperarsi per prevedere sgravi fiscali per le aziende che assumono personale residente in quei territori perché, anche in questo caso, o noi attuiamo politiche attive di lavoro e di sviluppo economico sui territori Grazie, in esame, in quanto esperienze similari hanno dimostrato che quando lo Stato crea sgravi e incentivi forti per le aziende che assumono, la curva delle assunzioni e dei contratti sale, mentre inevitabilmente scende quando questi finiscono (si veda la storia del *jobs In questo momento si tratta di una misura assolutamente essenziale per creare un volano di ripartenza dell'economia di questi territori, per garantire sviluppo e per dare lavoro ai cittadini che resistono in territori che non offrono più alcuna opportunità.

del 1° luglio 2018, previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che introduce nuove modalità di pagamento degli stipendi dei lavoratori tramite conto corrente bancario o postale. È evidente che ciò penalizza in particolare il lavoro con oneri economici maggiori sia per i lavoratori, che per i datori di lavoro in un territorio che già richiede e richiederà sforzi economici alle popolazioni. Fatta salva la sacrosanta tracciabilità delle somme corrisposte (che, ricordo, sarebbe garantita dal ripristino del *voucher*), chiediamo che il Governo si impegni a valutare l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2018 l'entrata in vigore della legge succitata o, quanto meno, fino al ripristino del *voucher*

in possesso delle amministrazioni e del Commissario per la ricostruzione, quindi fondi già disponibili, possano essere impiegati per reclutare personale anche attingendo, quando Grazie, società controllate *in* *house providing*. Di fatto, quindi, non c'è alcun aggravio di spesa, questa è una norma di buon senso che serve a mettere in condizione le amministrazioni comunali di poter attingere a personale che altrimenti ha forte difficoltà a reclutare e senza questo personale le pratiche non vanno avanti. Questo, tra l'altro, è un momento in cui la curva sta salendo perché, dopo tanto immobilismo e comunque tante difficoltà, la macchina della ricostruzione si sta mettendo in moto, il numero delle pratiche si moltiplica per dieci o per cento di giorno in giorno e se non arriva il personale, anche tecnicamente competente, in grado di lavorare le pratiche, la ricostruzione si blocca per ragioni banalissime. Invito banalissime. Invito il relatore e il Governo a rivedere la loro posizione di contrarietà, perché - ripeto - non c'è alcun aggravio di spesa, è una norma di buon senso che aiuta e semplifica la procedura e noi la stiamo proponendo in uno spirito assolutamente costruttivo e collaborativo per migliorare il testo

riguarda l'introduzione di una deroga al codice della strada per gli immobili risultati distrutti a seguito del sisma e vicini alle strade. Con questa norma se ne consentirà la perfetta ricostruzione,

quest'Assemblea e soprattutto le forze di opposizione hanno deciso di segnare un punto politico e noi abbiamo aderito a questo punto politico. E qual è il punto politico?

e proprio perché è arrivato alla scadenza - che sembrava l'ultima scadenza prima che si formasse il Governo - il decreto-legge in esame ha fatto lo stretto necessario, per rispetto delle forze politiche che poi avrebbero potuto scegliere altre priorità, che non quelle che chiediamo adesso di inserire nel decreto-legge, per arricchirlo con tutte le questioni che sono state anche sollevate dal territorio. Per tutte queste ragioni riteniamo di sottolineare che è una scelta politica il non aver trovato i soldi per coprire spese aggiuntive, perché dal primo minuto in cui si è in carica si assumono scelte politiche e che, più in generale, l'atteggiamento tenuto oggi dall'Assemblea *(Commenti del senatore

il Consiglio europeo fissato per domani e dopodomani costituisce un appuntamento molto importante per il futuro dell'Unione europea. Sono iscritti nell'agenda alcuni temi fondamentali come la migrazione, la sicurezza e la difesa europea, l'innovazione e il digitale, il lavoro, la crescita e la competitività, l'unione bancaria e monetaria e il prossimo quadro finanziario pluriennale, Grazie, come ho già precisato alla Camera - di rispondere alle aspettative reali dei cittadini con proposte concrete e con l'indicazione chiara di un percorso da seguire e di obiettivi da raggiungere, senza tentennamenti, senza ambiguità e senza paura. Mi riferisco a questo atteggiamento, a questa determinazione, quando parlo di quel cambiamento, nel metodo e nella sostanza, che ho annunciato dinanzi alle Camere e che, dal primo giorno di questo Governo, mi sono impegnato a proporre in tutti i contesti internazionali con la forza e la consapevolezza di un Governo che in Europa parla con una voce sola, ferma e risoluta. L'Italia, con il suo apporto sui vari temi, in special modo in tema di immigrazione, può contribuire a rendere questo appuntamento uno spartiacque, un punto di svolta e di cambiamento per l'Europa, in modo da contribuire a disegnare l'Europa che vogliamo e che intendiamo realizzare nel futuro prossimo venturo. In tema di immigrazione abbiamo ben presenti alcuni obiettivi, per i quali stiamo lavorando da tempo con la massima concentrazione. E, solo quando li avremo raggiunti, potremo rivendicarli e potremo dirci soddisfatti, non per noi, ma per ciò che questi obiettivi rappresentano di buono e produrranno nella vita degli italiani e anche in quella dei tanti migranti che oggi si avventurano in mare e sfidano la sorte, alla ricerca di un futuro migliore e invece rimediano morte, pericoli vari, frustrazione ed emarginazione. Come avrete saputo, abbiamo elaborato una proposta, che ho anticipato domenica scorsa a Bruxelles nell'ambito del prevertice, di un *summit* organizzato in vista della preparazione del Consiglio europeo: è una proposta che mira a offrire una regolamentazione puntuale e una gestione efficiente dei flussi migratori, anche dal punto di vista dell'interesse del nostro Paese e dei nostri cittadini. Siamo riusciti a far accantonare una bozza di proposta circolata anticipatamente, che risultava chiaramente inadeguata a offrire un'efficace soluzione al problema dell'immigrazione. Era una bozza che andava anche contro gli interessi del nostro Paese. Per questa via, ottenendo il ritiro di detto testo, l'Italia ha avuto un riconoscimento e si è ritagliata un ruolo significativo. È un primo passo, ma costituisce senz'altro un buon punto di partenza per il Consiglio europeo che ci attende. La questione per noi davvero importante, dirimente, è risolvere efficacemente il problema dei cosiddetti movimenti primari. Risolvere questo problema significa automaticamente operare una drastica riduzione dei movimenti secondari, che pure - come sapete - in questa fase e nell'attuale momento storico, preoccupano particolarmente alcuni nostri *partner* europei. Ciò che proponiamo è una *European multilevel strategy for migration*: una proposta articolata, organica, basata su un nuovo approccio, che consenta all'Europa di uscire da una gestione intesa in base a una logica emergenziale e di entrare, invece, in una nuova dimensione, che prevede una gestione basata su una logica strutturale, da riconoscere definitivamente come priorità dell'Unione europea. Abbiamo individuato dieci obiettivi, che in parte sono stati anticipati dai *mass media* e che voglio qui riassumere rapidamente. Primo obiettivo: intensificare gli accordi e i rapporti tra Unione europea e Paesi terzi, secondo una direzione che viene già direzione che viene già percorsa, da cui partono e transitano i migranti, e investire in progetti di sviluppo, di formazione e di occupazione, che contribuiscano a ridurre all'origine il fenomeno dell'emigrazione, prevenendo i flussi e, quindi, riducendo i viaggi della morte. Penso - ad esempio - a un'intensificazione dei rapporti con la Libia e il Niger, col cui aiuto abbiamo già ridotto in misura significativa le partenze nel corrente anno. Abbiamo il dovere concreto di prevenire che la vita e l'incolumità delle persone siano messe a rischio; un rischio che inizia ben prima che i migranti comincino l'attraversamento per mare e giungano alle frontiere terrestri europee. La solidarietà europea deve manifestarsi già in questa fase, in modo da tutelare efficacemente sia i diritti dei migranti, sia, nel contempo, la sicurezza dei nostri cittadini. Secondo obiettivo: creare centri di protezione internazionale nei Paesi di transito, per offrire assistenza e consulenza giuridica ai migranti stessi, in modo da gestire in via anticipata e rapida le richieste di asilo e organizzare i rimpatri volontari assistiti verso i Paesi di origine. Chiaramente una grande importanza rivestono in questa prospettiva i rapporti, peraltro già in corso, tra Unione europea e organizzazioni come l'Alto commissariato ONU per i rifugiati o l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Occorre stanziare ulteriori fondi, fondi più cospicui per il *Trust fund* dell'Unione europea per l'Africa; in particolare, la finestra del Nord Africa deve essere rifinanziata in modo cospicuo. Terzo rafforzare le frontiere esterne dell'Unione europea, con operazioni della stessa Unione europea, ma anche con il supporto della Guardia costiera libica, anche stipulando ulteriori accordi, oltre a quelli già esistenti, con Paesi nordafricani e mediorientali, volti se del caso a esternalizzare i controlli di frontiera, integrandoli anche con personale dell'Unione europea. Anche in questo caso vi sono missioni in corso, operation Sophia e Joint Operation Themis, che stanno già supportando efficacemente la Guardia costiera libica. Quarto che ritengo cruciale: occorre superare il regolamento di Dublino, che non va riformato, ma appunto superato perché del tutto inadeguato a gestire il problema dei flussi migratori. va detto anche alla luce dei dati statistici: sono circa il 7 per cento gli aventi diritto allo *status* di rifugiato. L'attuale sistema comune europeo di asilo si fonda su un tragico paradosso: i diritti delle persone che intendono richiedere asilo vengono riconosciuti soltanto nel momento in cui gli interessati riescono a raggiungere le coste dell'Europa. Questo momento va anticipato, anche al fine di tutelare i loro interessi e di garantire più sicurezza al nostro Paese.

Quinto obiettivo: va superato il criterio del Paese di primo arrivo. Anche questo non è un criterio idoneo per gestire i flussi in modo efficace e sostenibile. Va, infatti, affermato il principio - l'ho ripetuto con vigore in tutti gli incontri che ho avuto con i *leader* europei, in Francia con Macron e a Berlino con la Merkel - che chi sbarca in Italia sbarca in Europa. *(Applausi

- come tutti diciamo a parole - allora il criterio del Paese di primo arrivo va superato. Sesto obiettivo: l'Unione europea e gli Stati membri devono assumere una responsabilità comune europea sulle persone, gli uomini, le donne e i bambini salvati in mare. È impensabile che la responsabilità in ordine alle richieste di asilo ricada esclusivamente sul Paese di primo arrivo. Occorre superare il concetto di «attraversamento illegale» per le persone soccorse in acque internazionali. Quindi, occorre rivedere anche la disciplina delle attività di *search and rescue*. Bisogna, insomma, scindere il piano dell'individuazione del porto sicuro di sbarco dal piano dell'individuazione dello Stato competente a esaminare le richieste di asilo. L'obbligo di salvataggio, in accordo con il diritto del mare e le convenzioni internazionali, non può diventare obbligo di processare tutte le domande per conto di tutti. Settimo obiettivo: l'Unione europea deve contrastare con iniziative comuni ben più efficaci del passato la tratta di esseri umani *(Applausi e combattere più efficacemente le organizzazioni criminali che alimentano i traffici e le false illusioni dei migranti. Ottavo non possiamo portare tutti in Italia o in Spagna; occorrono centri di accoglienza in più Paesi europei per salvaguardare i diritti di chi arriva ed evitare ovviamente, al contempo, problemi di ordine pubblico e di sovraffollamento. Occorre poi che, nel quadro di ripartizione delle responsabilità, vengano realmente portati a termine i cosiddetti ricollocamenti e rinforzare i meccanismi e le modalità di rimpatrio al fine di rendere i rimpatri più effettivi. Nono obiettivo: occorre ovviamente prestare attenzione - come ci viene chiesto - ai movimenti secondari. È un problema che non possiamo trascurare. È certo che, attuando per bene i principi e realizzando gli obiettivi appena sopra esposti, gli spostamenti intraeuropei di rifugiati risulteranno marginali e potrebbero agevolmente diventare oggetto di intese tecniche tra i Paesi maggiormente interessati. Decimo obiettivo: ogni Stato - voi sapete - stabilisce quote di ingresso dei migranti economici. Questa è una facoltà riservata agli Stati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 75, comma Dobbiamo rispettare questa facoltà, anche perché non mi sembra questo il tempo di proporre cessioni di sovranità agli Stati in ordine alle politiche pubbliche sulla gestione dei flussi migratori. Questo principio, tuttavia, va controbilanciato con la previsione del rafforzamento di adeguate contromisure finanziarie nei confronti degli Stati che non si offrono di accogliere rifugiati. Nei miei contatti di questi giorni e delle ultime settimane con i *leader* europei, sto ripetendo un concetto semplice, che per noi è il cardine della strategia che abbiamo elaborato: per avere un'Europa più forte, abbiamo bisogno di un'Europa più giusta e più equa. Sulla migrazione sono in gioco i valori dell'Europa unita e l'Italia - lo dico con orgoglio, da Presidente del Consiglio di un grande Paese, fondatore dell'Unione europea - continuerà a fare la sua parte perché l'Europa sia all'altezza del suo compito. C'è in questo impegno italiano una coerenza con l'azione che, da sempre, il nostro Paese sta perseguendo: penso, in particolare, a quanto hanno fatto e continuano a fare le Forze armate, *in primis* la Marina militare, la Guardia costiera, i sindaci, i volontari; insomma, un intero e complesso sistema, tutto italiano, che da anni salva l'onore dell'Europa nel Mediterraneo.

Passando al tema del quadro finanziario pluriennale, anche in questo caso dobbiamo ribadire la necessità di avere un'Unione europea più giusta e più equa. Sono stati diffusi i dati Istat sulla povertà in Italia: non può essere ignorato che, nel 2017, oltre 5 milioni 5 milioni di persone in Italia hanno vissuto sotto la soglia della povertà assoluta. Stiamo parlando di un milione e 778.000 famiglie, di un aumento rispetto al 2016 che riguarda soprattutto il Meridione, nel quale l'incidenza della povertà assoluta è salita dall'8,5 per cento del 2016 al 10,3 per cento del 2017. Questi dati ci obbligano a dare risposte concrete: ci sono 5 milioni di persone che non possono più aspettare. Il problema della povertà si intreccia, poi, con quello del divario territoriale, anche questo intriso di ingiustizie e paradossi. Per questo, pretenderemo che l'Unione europea contribuisca a offrire risposte in entrambe le direzioni, consentendo un più ampio e organico utilizzo dei fondi strutturali dedicati a questi temi. Nel nostro programma di Governo abbiamo messo nero su bianco l'impegno per il lavoro e il reddito di cittadinanza per migliorare l'inclusione sociale e le opportunità di impiego, specialmente per i giovani, ma non solo. Nella discussione sul prossimo bilancio pluriennale, proporrò che il negoziato riservi un'attenzione finanziaria più sostanziale ai fondi dell'Unione europea a sostegno dell'inclusione sociale. Penso, in particolare, al Fondo sociale europeo, che potrebbe servire per finanziare - ad esempio - la riforma e il potenziamento dei centri per l'impiego, che sono il cardine della nostra proposta sul reddito di cittadinanza. Il bilancio 2021-2027 è uno strumento chiave per raggiungere questo traguardo, insieme allo scopo, fissato dalla Commissione, di un - cito testualmente - «bilancio moderno per un'Unione che protegge, rende più forti e difende». Per questo, il bilancio dell'Unione dovrebbe concentrarsi sui modi per sostenere la crescita nazionale e affrontare le sfide comuni in modo efficace. L'Italia è un contributore netto al bilancio dell'Unione. Pensiamo perciò di meritare una maggiore attenzione ai nostri bisogni anche per quel che riguarda specificamente le politiche tradizionali - penso all'agricoltura, alla coesione - e una risposta comune al fenomeno migratorio. Naturalmente, ci opporremo a qualsiasi misura che danneggi le Regioni e i territori ancora in difficoltà. Equità significa anche questo. Dirò che, in linea di principio, a concentrarci sulle nuove priorità di bilancio: migrazione e controllo delle frontiere, difesa e sicurezza, crescita e innovazione. Ma abbiamo bisogno di un aiuto più consistente e di espressioni di maggiore solidarietà da parte dell'Unione europea e di tutti gli Stati membri, per tutte le modalità che ho espresso. Veniamo ai temi del lavoro, della crescita, della competitività e dell'inclusione sociale, in parte già anticipati. Anche questi temi vanno affrontati con maggiore vigore e incisività da parte dell'Unione. Oltre al *focus* sull'occupazione e l'inclusione sociale nel bilancio settennale, il Consiglio si occuperà anche di misure per la crescita e la competitività. Intendiamo portare a Bruxelles la nostra visione sulla riforma del sistema tributario, spiegarla e contribuire al dibattito in quella sede. L'Italia ha bisogno di ridurre la pressione fiscale - come ci siamo impegnati a fare con il nostro programma di Governo e di accompagnare a questa misura la riduzione del cosiddetto *red tape*: la burocrazia che, unita alla pressione fiscale, ha conseguenze nefaste sulla qualità del rapporto tributario tra lo Stato e i contribuenti, come pure sulla competitività del nostro Paese. Il Consiglio europeo discuterà, dunque, anche di questa leva necessaria per rendere l'Europa più competitiva. appoggeremo tutti gli sforzi contro l'elusione e l'evasione fiscale. Cercheremo, in particolare, di progredire nella messa a punto di un sistema di definizione della base imponibile, superando la frammentazione dei sistemi di imposizione nazionali. Abbiamo bisogno di una Europa più equa anche a livello fiscale. L'attuale assetto europeo non garantisce una tassazione equa, per quanto riguarda - ad esempio - le attività dell'industria del *web*, le cosiddette *digital company*. Sosterremo un approccio deciso sulla soluzione europea, nell'attesa di una soluzione che auspichiamo anche a livello globale, per tassare adeguatamente i profitti generati negli Stati membri e restituirne i benefici alle comunità che hanno contribuito Infine, lavoreremo per ottenere soluzioni eque ed efficaci volte a risolvere le conseguenze negative generate dell'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein.

del mio discorso per la fiducia, che il nostro obiettivo è e resta l'eliminazione del divario di crescita tra l'Italia e l'Unione europea, e lo stiamo perseguendo in un quadro di stabilità finanziaria e di fiducia dei mercati. Il debito pubblico italiano è oggi pienamente sostenibile. Dobbiamo certamente puntare alla sua riduzione, ma in una prospettiva di crescita economica, e orienteremo la politica fiscale e di spesa pubblica al perseguimento degli obiettivi di crescita stabile e sostenibile. Questo è il nostro messaggio chiave in sede di discussione sulla *governance* economica della nostra Europa al prossimo Euro Summit del 29 giugno, a margine del Consiglio europeo. Resto ottimista sull'esito della riflessione che ci attende a Bruxelles, ma sarò molto chiaro sulle nostre posizioni: se vogliamo impedire il declino dell'Unione e realizzare una Unione in campo economico che sia percepita come realmente vicina ai nostri cittadini, è il momento di far avanzare la condivisione del rischio finora rimasta troppo indietro. Però, attenzione: questi meccanismi di condivisione del rischio non debbono contemplare condizionalità - per dirla nel gergo dell'Unione - che, in nome dell'obiettivo della riduzione del rischio, finiscano per irrigidire processi già processi già naturalmente avviati e in corso, con il risultato di ottenere, anziché la riduzione del rischio, l'incremento dell'instabilità bancaria e finanziaria non tanto non tanto in Italia, ma semmai in altri Stati membri caratterizzati da sistemi economici di più modesta entità e, quindi, più esposti. Per essere chiari, non vogliamo un Fondo monetario europeo che, lungi dall'operare con finalità perequative, finisca per costringere alcuni Paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti e automatici, con sostanziale esautorazione del potere di elaborare in autonomia politiche economiche efficaci. Siamo contrari a ogni rigidità nella riforma del meccanismo europeo di stabilità, soprattutto perché nuovi vincoli al processo di ristrutturazione del debito potrebbero contribuire essi stessi all'instabilità finanziaria, anziché prevenirla. Non vogliamo inoltre pericolose duplicazioni con i compiti della Commissione europea per la sorveglianza fiscale, che rischierebbero peraltro di delegittimare la base democratica di queste funzioni essenziali per la stabilità finanziaria. Passo ora alla materia Anche qui i progressi dell'integrazione europea sono stati significativi, particolarmente nell'ultimo anno e mezzo. Da parte nostra siamo a favore delle misure e degli strumenti di cooperazione tra gli Stati membri per evitare duplicazioni e dispersione delle spese: dalla difesa alla cooperazione strutturale permanente - la cosiddetta PESCO - che riunisce 25 Paesi dell'Unione europea in una cornice politica e giuridica di impegno comune per la difesa, al Fondo europeo per la difesa, dove si punta a raggiungere un accordo per la componente industriale. Tutte queste iniziative si completano e si rafforzano nell'ambito delle attività della NATO, alle quali l'Unione europea resta strettamente legata, così come il nostro Paese. Sempre nel quadro della cooperazione tra Unione europea e NATO, prosegue la riflessione per migliorare la mobilità militare, facilitando la circolazione delle forze militari all'interno dei confini europei per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Stiamo proseguendo anche sulla politica europea nel settore della sicurezza civile, essenzialmente attraverso missioni di rafforzamento delle capacità di selezionati Paesi terzi in materia di polizia e amministrazione civile e giudiziaria. Questo cammino proseguirà nei prossimi mesi e ne riparleremo in autunno. In materia di innovazione e digitale, i negoziati sul prossimo bilancio settennale saranno anch'essi cruciali per perseguire i nostri obiettivi di occupazione e crescita. Dobbiamo infatti assicurare che, nel prossimo quadro finanziario pluriennale, l'impulso europeo all'innovazione sia rivolto alla crescita e all'occupazione. Per fare questo, le regole europee devono incentivare e non scoraggiare gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo e gli stessi investimenti delle banche nell'innovazione. Lavoreremo a un approccio equilibrato all'innovazione, capace di incentivare quella di rottura, senza trascurare quella incrementale. In questo quadro, sosterremo un approccio dal basso che tenga conto delle esigenze delle imprese e le aiuti a creare nuovi posti di lavoro. Al Consiglio europeo ci sarà anche una discussione sull'attuazione degli accordi di Minsk, che - come sapete - è un dibattito importante rispetto alle sanzioni settoriali nei confronti della Russia. Su questo riaffermiamo il principio per cui non deve esserci nulla di automatico nel rinnovo delle sanzioni. Sul punto occorre molta cautela - ce ne rendiamo conto - ma la nostra impostazione muove dal principio cui le sanzioni sono un mezzo e non un fine. Continueremo, quindi, a dare grande attenzione al sostegno alla società civile russa e anche agli interessi delle nostre imprese, piccole e medie. una considerazione finale sul tema della Brexit. La questione più difficile su questo versante resta quella del confine tra Irlanda e Nord Irlanda, su cui continueremo a lavorare nelle prossime settimane, con l'obiettivo di preservare la pace e l'Accordo del Venerdì Santo ed evitare la sciagurata ipotesi di un recesso senza accordo, che sarebbe inaccettabile anche per le imprese e i cittadini. Anche per questo motivo porterò all'attenzione dei miei colleghi europei la difesa senza ambiguità dei diritti dei nostri connazionali che vivono nel Regno Unito per avere dalle autorità britanniche impegni precisi e puntuali, vigilando in particolare sui diritti delle categorie più vulnerabili e in difficoltà. Si negozia l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ma, nello stesso tempo, dobbiamo costruire per il futuro un partenariato che rifletta il profondo legame tra la Gran Bretagna e il continente europeo. L'Italia, in particolare, lavorerà per un partenariato basato sulla mobilità, per garantire che i fruttuosi scambi tra i nostri cittadini possano continuare; sull'economia per mantenere un elevato scambio dei commerci e sulla sicurezza per affrontare insieme in maniera più efficace le numerose sfide del nostro tempo. Vi ringrazio per l'attenzione.

ma, soprattutto, la ringrazio per il lavoro che sta portando avanti per tutelare noi cittadini. A nostro avviso, lei ha agito nel migliore dei modi ed io, per la prima volta, mi sento davvero rappresentata in Italia, in Europa e all'estero. La Il tema dell'immigrazione e della *governance* economica dell'Unione europea saranno al centro del prossimo Consiglio europeo. In questi ultimi giorni, non ho potuto fare a meno di notare quanto sia complicato parlare di questi temi, in un contesto in cui gli interessi economici sono più importanti del benessere delle persone. Sull'immigrazione è arrivato il momento di voltare pagina. È necessario trovare delle soluzioni comuni perché, senza un rafforzamento della gestione europea, il fenomeno migratorio non può essere governato ed è destinato a rimanere senza controllo. L'Unione europea dovrà rafforzare i rapporti con i Paesi di origine e di transito dei migranti, così da prevenire i viaggi della morte. morte. Cari colleghi, sebbene alcuni di voi ci abbiano accusato di essere cinici e imprudenti, il valore che più abbiamo a cuore è la salvaguardia della vita umana. Per questo, il nuovo approccio al fenomeno dell'immigrazione sarà orientato a tutelare i diritti fondamentali dell'uomo, dichiarando una guerra senza precedenti a tutti i trafficanti di esseri umani. Quello che auspico è che questa guerra non venga combattuta soltanto dall'Italia, com'è accaduto negli ultimi anni. Siamo rimasti soli davanti a questa emergenza, ma credo che un cambio di paradigma nella gestione dell'immigrazione giovi non soltanto all'Italia, ma anche al resto dell'Europa. Agire insieme rafforzerà i vincoli di solidarietà tra gli Stati, perché un'Europa dove c'è un Paese che traina e Paesi che vengono trainati non è un'Europa che funziona. Caro Presidente, l'Italia è stata relegata a una condizione di subalternità anche in altri ambiti. A questo proposito, vorrei sottoporre alla sua attenzione alcune questioni relative alla riforma dell'unione economica e monetaria, anzitutto la modalità attraverso cui il Meccanismo di vigilanza unico monitora lo stato di salute delle banche. Questo sistema di valutazione si è concentrato prevalentemente sul rischio di credito, trascurando il rischio di mercato relativo alla presenza nei bilanci bancari di strumenti finanziari derivati. Questo meccanismo ha determinato uno svantaggio per i sistemi bancari più focalizzati nella tradizionale attività creditizia, come ad esempio quello italiano, avvantaggiando, invece, i sistemi bancari maggiormente orientati alla speculazione finanziaria, come quelli francesi e tedeschi. Come sappiamo, l'unione bancaria è ancora priva del suo terzo pilastro, cioè il Sistema europeo di assicurazione dei depositi, l'EDIS. Alcuni Paesi ritengono che le banche degli Stati membri potranno condividere i propri rischi tramite l'EDIS solo dopo averli drasticamente ridotti. L'idea di ridurre i rischi prima dell'istituzione dell'EDIS è condivisibile, ma a condizione che si considerino tutti i rischi e non solo alcuni. Infatti, se i crediti deteriorati se i crediti deteriorati e i titoli di Stato possono costituire una fonte di rischio per le banche tradizionali, per altre banche rischi rilevanti scaturiscono dal possesso di strumenti finanziari derivati. Nel 2016 le attività e le passività di livello 2 e livello 3 detenute dalle maggiori banche europee ammontavano complessivamente a 6.800 miliardi di euro, un valore circa 12 volte a quello dei crediti deteriorati di tutte le banche dell'area dell'euro. Caro Presidente, lavoriamo insieme e noi saremo sempre al suo fianco per una Europa più equa. *(Applausi

Pertanto, vorremmo sapere da lei qual è la visione complessiva sulle relazioni internazionali, sulla politica internazionale e comunitaria del nostro Paese; qual è la cornice. Rimaniamo in un ambito multilaterale o si privilegia essenzialmente il canale bilaterale? Ancora, con quali alleanze? Lo dico perché i successi che abbiamo ottenuto con la nostra diplomazia e con i nostri Governi negli anni passati li abbiamo raggiunti costruendo delle alleanze solide. È stato così sui flussi migratori, con il passaggio da Triton a Themis, l'operazione Sophia, la modifica di Frontex e la maggiore attenzione sul Mediterraneo; L'abbiamo fatto costruendo delle alleanze. Anche riguardo al proposito giusto di modificare Dublino (peraltro approvato con il supporto di una forza politica che oggi sostiene tale proposito), noi condividiamo l'idea, invece, di superarlo, PD)*. Ma con quali alleanze? Con i Paesi di Visegràd o con quelli con cui noi stiamo provando a costruire, giustamente, un cordone positivo nel Mediterraneo? E questo vale anche per il Sud della Libia e il Niger. Abbiamo sentito le parole di Salvini di ritorno dalla Libia. Ebbene, io consiglierei più prudenza. prudenza. I Ministri che si sono susseguiti hanno usato prudenza quando tornavano dalla Libia. A proposito del Sud della Libia e del Niger, io vorrei ricordare che i Governi precedenti hanno aperto l'ambasciata in Niger. Hanno avviato la costruzione di una missione, quella stessa missione alla quale le forze politiche che la sostengono hanno detto di no, perché era un intervento coloniale. Mi fa piacere adesso sentire Salvini dire che dobbiamo concentrare lì le nostre attenzioni. *(Applausi dal Gruppo d'emergenza per l'Africa, che va rafforzato. Noi siamo stati i primi a destinarvi dei soldi, perché lo *slogan* "aiutiamoli a casa loro" non deve essere usato solo in campagna elettorale. Poi bisogna essere conseguenti e portarlo avanti con provvedimenti concreti. Ci fa piacere, dunque, che lei vada in questo senso. Dico ciò, più in generale, sulla visione di politica estera. Voglio dire che i nostri punti cardinali sono stati tenuti come una barra dritta dai Governi che si sono succeduti, anche di colore diverso. Qui ci siamo confrontati con sensibilità e declinandoli in maniera diversa, ma sono stati chiari: la scelta atlantica come un insieme di valori prima ancora che come scelta che garantisse la sicurezza e la stabilità del nostro continente; la scelta europea la scelta europea e la costruzione europea come modo per evitare gli egoismi nazionali e garantire un futuro al nostro Paese; affrontare quelle scelte che non si è più in grado di affrontare con mere misure nazionali. E, infine, l'equilibrio nel Mediterraneo e nel vicino Oriente, dove abbiamo declinato responsabilità e solidarietà; dove non siamo andati a bombardare ma abbiamo fatto operazioni di *peacekeeping* e dove siamo andati a costruire e ricostruire le istituzioni. *(Applausi Sì, abbiamo salvato vite, perché il tema della responsabilità e della solidarietà vanno di pari passo. E, se noi abbiamo garantito la stabilità e la sicurezza nel nostro Paese, è perché abbiamo seguito quella strategia. Quindi, società aperta, stabilità e sicurezza vanno avanti di pari passo con una politica estera chiara che tenga saldo il timone. Lo dico perché questo equilibrio delicato non è per sempre; è una conquista faticosa di ogni giorno ed è lì che si misura la differenza tra la propaganda e la politica. Buon lavoro. Signor Presidente del Consiglio, nel suo discorso, che ho ascoltato - un discorso articolato e complesso

La storia ci ha raccontato a lungo di un sogno utopico, di un futuro prospero - perché ce lo chiedeva l'Europa e di Stati cattivi perché sovrani. Questa storia non regge più. Le popolazioni europee chiedono risposte e gli italiani pretendono risposte. È giunto il momento di un nuovo inizio e il Consiglio europeo che parte domani deve dare un segnale; non c'è più tempo. ha sviluppato diversi punti. Io mi soffermerò solo su alcuni dei temi che lei ha trattato. Prima fra tutte c'è la questione dei migranti, che coinvolge il nostro Paese e tocca un nostro ex alleato, il nostro principale alleato nel continente africano, la Libia.

delle politiche del Governo, queste cose le deve dire. La Libia era il primo alleato dell'Italia nel continente africano. La caduta di quel Governo o di quel regime, comunque lo si voglia chiamare, è stata un danno soprattutto per il nostro Paese, mentre è stata un vantaggio innegabile in particolare per alcuni dei nostri alleati, che sono alleati all'interno della NATO,

un Paese ormai completamente destabilizzato e dal quale partono quasi tutti i flussi migratori. Oggi la Francia cerca il controllo della Cirenaica e cerca di arrivare probabilmente a controllare anche la Tripolitania. allora forse auspicabile che le politiche del Governo in tema di cooperazione e sviluppo in quel Paese riprendessero a trattare le cose semplici che caratterizzavano la presenza italiana in Libia, con le persone che partivano dall'Italia settimanalmente e andavano a fare i lavori comuni, perché quella era la reale presenza italiana, quella delle piccole e medie imprese, come delle grandi imprese italiane che, non solo avevano fatto crescere e costituito nuovamente

provare a ricostruire quel tessuto connettivo con il nostro contributo, facendo anche, in un certo senso, la voce grossa con i nostri alleati nell'Unione europea e nella NATO, ricordando che non è più possibile possibile che il nostro Paese continui a considerare azioni fatte a nostro discapito e a beneficio di altri come la linea da seguire nei prossimi anni.

Il 28 e il 29 giugno si cercherà infatti di capire se un'organizzazione, che negli anni si è trasformata in un insieme di indifferenze, ipocrisie e sofferenze, possa tornare a considerarsi una comunità

come un Paese libero, sovrano e indipendente, con una politica estera che abbia soprattutto a cuore gli interessi strategici nazionali. Solo così, per l'Italia in primo luogo, ma anche, in secondo luogo, per il resto dell'Europa, potrà esserci un futuro e potranno esserci gli strumenti per affrontare in modo credibile le sfide del domani. ancora, l'immigrazione, credo sia il momento di ribadire con grande forza che le politiche dei Paesi occidentali, tese spesso e volentieri a mantenere il possesso e la gestione delle materie prime in Africa e in Medio Oriente, siano state volano di destabilizzazione e *caos*. A milioni si contano i morti, tra profughi e disperati: chi è responsabile? Vorrei concludere con una notazione che considera le parole del presidente Macron, del presidente Macron, il quale ha detto, qualche giorno fa, che non si possono avere Paesi che beneficiano largamente della solidarietà dell'Unione europea e allo stesso tempo mostrano egoismo quando si parla dei migranti. Sappiamo a chi si riferiva, ma in questo caso ritengo che tali parole siano giuste. Il presidente Macron ha ragione: sì, il comportamento di Francia e Germania è stato davvero inaccettabile ed è il momento di porvi fine.

Presidente, colleghi, vorrei dire al presidente Conte, con molto rispetto, che non riusciamo ad essere soddisfatti per come il nostro Governo si è mosso in vista del prossimo Consiglio europeo. Un Governo che si dice "del cambiamento" dovrebbe attuare dei cambiamenti tangibili o, quantomeno, creare condizioni favorevoli all'attuazione di cambiamenti tangibili. Ebbene, di cambiamenti non ne abbiamo visti, o meglio ne abbiamo visti pochi e quelli che vediamo non sono positivi. Ci pare evidente che poco o niente sia stato fatto per arrivare a dei cambiamenti positivi. Nel campo della politica estera e di quella migratoria in particolare, le dichiarazioni di principio, le enunciazioni vaghe, alle volte fino ai confini della banalità, hanno un senso e una incisività solo se vengono seguite da risultati concreti. La domanda che dobbiamo porci è questa: stiamo ottenendo dei risultati concreti? Non ci pare. C'è stata un'innovazione di metodo - questo sì - ed è consistita in ciò: il Ministro dell'interno rompe tutto e poi, dopo alcuni giorni o alcune ore, il Presidente del Consiglio prova a riattaccare qualche coccio. È forse questa una sana divisione del lavoro? No, presidente Conte, me lo lasci dire. A parte che sui problemi decisivi non possono esserci nel Governo due voci e due linee - e men che meno tre o quattro voci e linee questo metodo del politico buono, che arriva a moderare gli eccessi del politico cattivo, rappresenta una garanzia di insuccesso, sulla scena nazionale e su quella internazionale *(Applausi dal Gruppo PD)* e rende la nostra azione internazionale

Possiamo dire di aver fatto passi avanti sul rafforzamento di Frontex e della protezione europea delle frontiere, sulle regole europee per l'asilo, sul superamento delle disparità contributive per gli arrivi che provengono dalla rotta mediterranea in confronto ai contributi che ci sono per gli arrivi che provengono dalla rotta balcanica? Possiamo dire di aver fatto passi avanti sui movimenti secondari, di averli fatti sulle sanzioni per i Paesi che non mostrano solidarietà? Su tutti questi fronti purtroppo finora nessun risultato è arrivato. L'unica cosa avvenuta è la seguente: Paese da una parte si è prestato all'accusa di realizzare colpi di mano propagandistici sulla pelle di persone inermi, chiudendo i porti a navi impegnate in attività di salvataggio, dall'altra ha acuito le tensioni con i Paesi a noi tradizionalmente più vicini e che erano e restano indispensabili per arrivare a modifiche migliorative del Regolamento di Dublino. Insomma, finora abbiamo visto una politica che combina alta visibilità, scarsa credibilità e assenza di realizzazioni concrete. È paradossale che si pensi di ottenere davvero qualcosa di tangibile sulle politiche di accoglienza, che hanno bisogno di più forti politiche sovranazionali e di condivisione degli oneri tra i vari Stati, facendo il filo all'Ungheria, alla Polonia, alla Repubblica Ceca, alla Slovacchia, al Vice *Premier* austriaco, al Ministro degli esteri tedesco. presidente Conte, avvertiamo la necessità di rivolgerle un suggerimento: incida di più sul modo di porsi del suo Governo. Finora l'Italia ha fatto notizia, più che per le proposte ragionevoli che avanzato, per le forzature scomposte che ha messo in campo. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Con la politica degli atti simbolici e delle spallate non si va da nessuna parte: si ottengono dei titoli ma non dei risultati. Come dimostra l'operato del Governo che ha preceduto il suo, si può essere allo stesso tempo umani a rigorosi, umani ed efficaci. *(Applausi dal Gruppo nella non invidiabile impresa di apparire allo stesso tempo poco umano e poco efficace; il suo Ministro dell'interno - ed è l'ultima cosa che dico - afferma che oggi siamo più forti e più rispettati, purtroppo non è vero: l'Italia è più debole e più isolata. Nei giorni scorsi un osservatore ha spiegato la situazione in termini chiari: pensare di conquistarsi la considerazione dei nostri *partner* dell'UE urlando di più è controproducente come cercare di farsi rispettare di più dai vicini di casa spingendo al massimo il volume del televisore. Signor Presidente del Consiglio, trovo che questa affermazione contenga una solida e chiara verità; gliela offro garbatamente, la ponderi, la soppesi, la valuti. Spesso alzando la voce si risulta solo più rumorosi, non più autorevoli, e se si ricorre di continuo alle esibizioni muscolari si finisce per apparire non più solidi ma solo più aggressivi. Come è stato suggerito da alcuni analisti, è saggio non anteporre l'ideologia all'interesse nazionale e comprendere che l'interesse nazionale lo si serve in maniera piena cercando in questa fase di essere protagonisti come Italia in un'Europa più forte e non facendo i Pierini in un'Europa più debole. Non è questo che secondo noi oggi serve all'Italia.

sulla base della proposta presentata dal presidente Jean Claude Junker all'Europarlamento lo scorso 2 maggio. Abbiamo preso atto di come l'iniziativa della Commissione persegua l'obiettivo di modernizzare il bilancio dell'Unione, rendendolo più flessibile (anche attraverso l'introduzione di strumenti speciali), semplice e trasparente, riducendo gli oneri burocratici per i beneficiari e prestando maggiore attenzione al valore aggiunto europeo degli interventi ammessi al sostegno dell'Unione. Il nuovo bilancio, basato su un rafforzamento del legame tra finanziamenti e rispetto dello stato di diritto, e su un approccio equilibrato nella gestione del disavanzo provocato dalla Brexit, sarà incentrato sulle priorità dell'Unione europea, così individuate: mercato unico; innovazione e agenda digitale; coesione e valori; risorse naturali e ambiente; migrazione e gestione delle frontiere; sicurezza e difesa, vicinato e resto del mondo e pubblica amministrazione europea. La Commissione propone, tra l'altro, di innalzare in modo significativo gli attuali livelli di finanziamento in settori quali la ricerca e l'innovazione, il sostegno ai giovani, l'economia digitale, la gestione delle frontiere, la sicurezza e la difesa, a fronte di una proposta di riduzione dei finanziamenti nei settori tradizionali della politica agricola comune e della politica di coesione. Sicurezza e difesa, dunque, con i seguenti tre settori. la protezione delle vittime di reati. Europol e azioni per la disattivazione nucleare in Lituania e la sicurezza nucleare e disattivazione in Bulgaria e Slovacchia. Difesa, Difesa, con il Fondo europeo per la difesa, che disporrà di 13 miliardi, dei quali 4,1 per il finanziamento della ricerca collaborativa e 8,9 a integrazione dei contributi nazionali per cofinanziare progetti collaborativi di sviluppo delle capacità e il meccanismo per collegare l'Europa, all'interno del quale una dotazione di 6,5 miliardi sarà riservata a potenziare le infrastrutture di trasporto, in modo da renderle idonee alla mobilità militare. Come non condividere, quindi, la sollecitazione del capo di stato maggiore della difesa, generale Claudio Graziano, quando afferma

Occorre insistere, quindi, secondo quanto da lei suggerito. Alle persone che continuano e si ostinano a rimanere miopi rispondiamo che occorre guardare con occhi che vogliono vedere e che credono in quello che vedono. E noi ci crediamo. Grazie, signor Presidente, e buon lavoro.

Signor Presidente del Consiglio, vorrei iniziare esprimendole gratitudine, la gratitudine che mi portano le persone che incontro per strada, le quali si sentono sollevate dal fatto che il Governo che lei guida stia restituendo al Paese un sano orgoglio patriottico, che è il migliore antidoto contro le derive del nazionalismo. Mentre organizzavo le idee per questo intervento in Aula, mi è capitato il foglio nel quale ho preso appunti quando lei è venuto a presentare il Governo. Mi era rimasta impressa una frase, che poi effettivamente ha fatto i titoli di tutti i giornali: sarò l'avvocato difensore del popolo italiano. E la domanda era: perché il popolo italiano dovrebbe aver bisogno di un avvocato difensore? Perché siamo perennemente sul banco degli accusati? Perché dobbiamo sentirci così in Europa? fondo i numeri, compresi alcuni dati che lei ha ricordato, segnalano che il nostro Paese, che è un Paese fondatore, è un contribuente netto a questo progetto. E questa cosa dobbiamo rivendicarla; già semplicemente rivendicare con forza e con autorevolezza questo semplice dato contribuisce a restituire al Paese il senso del proprio ruolo all'interno di questo progetto. Mi è venuto in mente, quando lei ha ricordato oggi questo fatto, un intervento su twitter di un collega di un'università tedesca, Sebastian Dullien, che il 5 giugno scorso si chiedeva si chiedeva quanti siano i tedeschi che sanno che in effetti l'Italia è un Paese contribuente netto. Le difficoltà che abbiamo incontrato nelle sedi europee sono dovute sostanzialmente a un racconto sbagliato del ruolo dell'Italia, sia in termini sia, più in generale, in termini politici, all'interno di questo progetto. Tale ruolo è sempre stato visto in termini negativi, e questo - mi duole dirlo non solo da parte dei *partner* europei, i quali naturalmente, nell'ambito di una normale dialettica in quella che è una Unione basata su una forte competizione, hanno l'interesse a descrivere come responsabili delle problematiche emerse soprattutto nell'ultimo decennio i Paesi del Sud (i cosiddetti PIGS). Purtroppo, al racconto di un'Italia perennemente sull'orlo del disastro hanno contribuito spesso anche le *élite* che questo Paese governavano, la retorica della perenne emergenza è stata uno strumento di governo; è stata il principale strumento attraverso il quale molti Governi che ci hanno preceduto hanno voluto

Quello che va apprezzato nella valorizzazione del Paese è proprio questa uscita dalla retorica dell'emergenza, dalla retorica del «fate del «fate presto», e questa volontà di costruire con ponderatezza un rapporto effettivo con l'Unione europea. Secondo quanto percepiamo e in base a quanto la popolazione intorno a noi percepisce, lei sta riuscendo con la sua squadra di Governo in questo scopo. Prima il collega Petrocelli si domandava a chi avessero giovato i bombardamenti della Libia, che è una domanda che tutti ci siamo posti

che, secondo uno studio di Rocholl e Stahmer del 2016, meno del 5 per cento dei soldi conferiti ai cosiddetti fondi di salvataggio nel caso della Grecia sono finiti effettivamente al Governo greco. Il 95 per cento dove è finito? *(Applausi Chi applaude sa la risposta, e a chi non applaude la do io: sono finiti a salvare le banche francesi e tedesche. Nulla di male in questo; non vogliamo la distruzione delle banche francesi e tedesche, ma vogliamo ridare un senso nuovo alla parola solidarietà. ricordo lo studio di Dany, Gropp, Littke e von Schweinitz dell'Istituto di economia di Halle del 2015. Quanto ha guadagnato la Germania dalla gestione della crisi? Nella gestione della crisi la Germania, in termini di riduzione di spese per interessi ha guadagnato oltre 100 miliardi. Come? Perché si è creato un meccanismo di fuga verso un Paese che veniva propagandato come sicuro, e anche perché si sono adottate delle politiche che erano fortemente tarate sull'interesse di quel Paese. Ora, in quel Paese che ci è stato propagandato come un porto sicuro per i soldi degli investitori europei, accade che ci sia una banca,

Grazie,

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi senatori, il Consiglio europeo di giovedì e venerdì vedrà al centro dell'agenda il tema delle migrazioni: un tema delicato su cui, più di ogni altro, si mettono in mostra le criticità di questa nostra Europa, si scontrano interessi e sensibilità diverse e su cui persino le tradizionali famiglie politiche europee si ritrovano su posizioni contrastanti. Tutto ciò mi porta a dire che, ben più dei timori smossi da alcune considerazioni sull'euro, forse è la posizione fragile di Schengen che dovrebbe preoccupare il futuro del nostro continente. Del resto, conscio di quanto sia dirimente la questione immigrazione, il presidente Juncker ha convocato un vertice informale domenica scorsa, iniziando così ad affrontare questa questione. E su tale questione si gioca davvero moltissimo, come ho già detto, della credibilità dell'Europa. In Italia abbiamo avuto di recente le elezioni - e qui lo sappiamo bene tutti sappiamo bene anche quanto la questione immigrazione abbia condizionato le scelte degli elettori italiani; era un tema che doveva essere sicuramente sdoganato, nessuno lo nasconde, perché è di primaria importanza. La presenza diffusa di centinaia di migliaia di migranti non integrati - e, ripeto, non integrati - molti dei quali irregolari (stime parlano di circa 600.000 irregolari, ovvero quelli che non finiscono nelle statistiche che spesso ci vengono mostrate anche da alcuni nostri colleghi europei) e la gestione inadeguata del fenomeno dell'accoglienza fanno percepire agli italiani un sentimento diffuso di insicurezza. poi la situazione economica: i recenti dati dell'ISTAT mostrano un Paese con 5 milioni di poveri e questo ci fa chiedere per quali ragioni si debbano utilizzare risorse pubbliche per sostenere un'accoglienza oltre le nostre possibilità. Ci fa anche chiedere perché non destinare quelle risorse a migliorare un sistema di inclusione imperfetto, perlomeno per come è congegnato, per i nostri poveri. Le somme messe a bilancio, infatti, mostrano appostamenti per quasi 5 miliardi di euro per gestire il fenomeno dell'accoglienza ai migranti. Tra l'altro sono somme - soldi degli italiani - che in buona parte sono state concesse come spesa in *deficit*; come dire che lasceremo i debiti ai nostri figli per sostenere l'accoglienza ai migranti. chiedo quali figli gli italiani avranno, vista la grave situazione occupazionale in cui versano i nostri giovani, la difficoltà a mettere su famiglia e il tasso di disoccupazione imbarazzante. Gran parte dei nostri studenti, formati nel nostro Paese, a spese del nostro Paese, sono, anche loro, costretti a fare un un viaggio, non in barca, ma comunque verso altri lidi. Noi di Forza Italia ci teniamo, invece, che cresca un altro tipo di disoccupazione: la disoccupazione degli scafisti e di chi, sulla pelle dei migranti e di persone in difficoltà, spesso va a lucrare. Dunque è curioso, perché investiamo solo 2 miliardi di euro destinandoli all'inclusione degli italiani. Non si tratta assolutamente di mettere poveri contro poveri o di inseguire politiche demagogiche, a volte urlate, ma di ragionare con coscienza sull'esistente, per migliorarlo nell'interesse dei nostri cittadini. Va detto, quindi, che resta un problema, che è quello dei nuovi sbarchi, che devono essere limitati proprio perché i nuovi arrivi andrebbero ad aggravare ulteriormente la situazione già pesante della gestione dell'accoglienza in Italia; un sistema di accoglienza che oggi si fa carico di poco meno di 200.000 persone, persone, con costi esageratamente alti; un sistema di accoglienza, inoltre, che ogni giorno sulla cronaca nera mostra non solo i suoi limiti, ma addirittura lo sconfinamento in gestioni che richiedono l'intervento della magistratura. Concedere 1.050 euro al mese per ogni adulto e 1.250 euro per ogni minore non accompagnato ha mosso gli appetiti della criminalità organizzata. Gli italiani riescono a vivere con molto meno e addirittura viene considerato povero un nucleo familiare di tre componenti che disponga di 1.044 euro al mese in alcune zone del Sud nel nostro Paese. La riduzione degli sbarchi, dunque, è prioritaria a ogni intervento. Il nostro sistema di accoglienza può smaltire le domande di asilo esistenti in un paio di anni solo se verranno fermati gli arrivi. Già ora il taglio delle domande di asilo ci dice che 60 domande su 100, come ci ha ricordato anche lei, non vengono accolte e a circa il 25 per cento delle domande viene concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si pone però un piccolo problema: il permesso per motivi umanitari deve essere abolito perché non trova applicazione negli altri Solo il 15 per cento delle domande di asilo accolte ha caratteristiche riconosciute in tutta Europa (rifugiato o protezione sussidiaria); la protezione umanitaria finisce per accogliere, quindi, migranti economici, che sono il primo motivo per cui l'Unione europea non accetta i ricollocamenti dell'Italia, fermi a 13.000 unità sulle 35.000 programmate. È una delle ragioni per cui i Paesi europei si preoccupano soprattutto di limitare le migrazioni secondarie. Se andiamo in Europa a negoziare un maggiore coinvolgimento dei *partner* europei nella gestione del fenomeno migratorio, dobbiamo quindi, innanzitutto, impegnarci ad abolire una una tipologia di protezione non prevista dall'Europa stessa. Signor Presidente, questa è una cosa che può fare questo Governo, perché fa parte del contratto di Governo e faceva parte anche del programma elettorale della coalizione di centrodestra. Noi di Forza Italia siamo da sempre stati capaci di critica, coraggio e, al contempo, atteggiamento propositivo nei confronti

il problema migranti chiama in causa, ovvero la capacità dell'Europa di prendere decisioni come soggetto politico unitario. Ad oggi ogni decisione è stata assunta dalla somma o sottrazione degli orientamenti dei singoli Stati. La invitiamo, quindi, ad adoperarsi per un'Europa che lavori davvero in modo unitario con concretezza

Signor Presidente, onorevoli senatori, Presidente del Consiglio, ho apprezzato le comunicazioni del presidente del Consiglio Conte in vista del vertice europeo. Non si tratta di parole di rito. L'Italia ha acquisito una centralità che da tempo non aveva nella politica europea. L'azione unitaria e decisa del nostro Governo e, forse, energica ha aperto un'evidente crepa nel muro di silenzio e di indifferenza che ha caratterizzato l'Europa in questi anni sulle vicende dei naufraghi e dei migranti. Se il Governo italiano non fosse stato risoluto, il problema sarebbe ancora oggi soltanto italiano e non avremmo ottenuto la disponibilità all'accoglienza di altri Paesi. La centralità italiana è stata annunciata dall'oggetto del mini vertice di domenica scorsa, nel quale si è sostanzialmente discusso soltanto della bozza presentata dal nostro Presidente del Consiglio e non di altri temi di maggior comodo per alcuni *partner* come i cosiddetti movimenti secondari. Fa un certo effetto la posizione dell'opposizione che nella scorsa legislatura, quando era maggioranza, nulla ha avuto da dire sulle condotte - chiamiamole disinvolte - del Governo Renzi. Non è un senatore 5 stelle a muovere queste osservazioni. La stessa senatrice Bonino, infatti, ha ricordato per ben due volte (nel luglio 2017 e, ancora, pochi giorni fa) che fu il Governo Renzi, tra il 2014 e il 2016, a proporre che gli sbarchi avvenissero tutti in Italia. La collega ha condivisibilmente parlato, al riguardo, di accordo scellerato. La Guardia costiera italiana avrebbe dovuto coordinare i soccorsi e gli sbarchi sarebbero dovuti avvenire in Italia. In cambio - cito ancora la collega Bonino - l'Italia avrebbe dovuto godere di maggiore flessibilità in termini di bilancio. È una posizione politica che condivido. Si è detto spesso che negli ultimi anni gli sbarchi dal Nord Africa fossero in calo, ma non si è mai parlato del costo umano di questo successo vantato all'ex ministro Minniti. L'Algeria ha ricevuto 111 milioni di euro per il contrasto alla partenza dei migranti. Dall'aprile del 2017 sono state abbandonate nel deserto del Sahara più di 13.000 persone, tra cui tantissime donne e bambini. Recentissimamente è emerso il crudele trattamento cui sono stati sottoposti alcuni migranti trattenuti nei campi libici negli ultimi anni: denutriti, picchiati, torturati e le donne stuprate. Se questo è il prezzo da pagare per far registrare un crollo degli sbarchi, non c'è certo da vantarsene. Nell'immobilismo ultraventennale appena perturbato da questi orridi compromessi era prevedibile che l'odierna risolutezza del Governo non fosse ben vista da coloro che erano abituati a un agire felpato o, diciamo, irrilevante. Ancora, mai nessuno nel Governo e nella maggioranza ha invocato l'arretramento della Guardia costiera. Posso dire che i miei - e li conosco bene - di certo non vogliono arretrare, sapendo bene che, se le motovedette sono opportunamente disposte nello scenario operativo, non solo le persone in difficoltà sono più tutelate, ma gli stessi equipaggi lavorano meglio e affrontano minori pericoli. Per quanto si tratti di scelte tattiche e operative, è chiaro che spetta alla politica nazionale ed europea assumersi tutte le responsabilità, poiché il complesso fenomeno formato dal soccorso in mare e dall'immigrazione non è ordinaria amministrazione. L'Italia non ha mai mancato di salvare e di soccorrere, ma quasi sempre è stata l'unica a intervenire. Non si sono quasi mai viste navi di altri Paesi. La nostra Guardia costiera ha svolto e svolge ancora oggi con onore una missione della quale dobbiamo andare fieri. È di queste ore la notizia di un incontro tra il Presidente del Consiglio italiano e il Presidente della Repubblica francese, nel quale si è individuato un principio generale sulla base del caso della nave Lifeline: superando i mortiferi accordi di Dublino, si è deciso che i naufraghi della Lifeline, ancorché sbarcati nel porto maltese de La Valletta, dovrebbero poi essere distribuiti tra i vari Paesi dell'Unione. La disponibilità all'accoglienza è già arrivata da Francia, Portogallo e Malta, oltre che dal nostro Paese, mentre stanno valutando ancora Spagna, Olanda e Germania. Indiscutibilmente si tratta di un successo del Governo. Anche la Commissione europea ha osservato che: «Non è giusto che sia solo un Paese dell'Ue a ricevere tutte queste navi e abbiamo compreso la posizione dell'Italia». Noi diciamo: finalmente!

Il ministro della difesa Trenta, coerentemente con l'azione unitaria del Governo, ha affermato - correttamente - che la sponda Sud è frontiera d'Europa e l'Unione ha il dovere di farsi carico della vigilanza e dell'immigrazione. Voglio concludere dicendo che tutti i Paesi dell'Unione dovranno assumersi le proprie responsabilità, e certamente non aiuta la posizione di chiusura del cosiddetto gruppo di Visegrád. Agli egoismi, alle miopie e ai piccoli calcoli effimeri dovrebbe conseguire una rivalutazione circa la sussistenza e la permanenza dei requisiti di democraticità per la permanenza nell'Unione europea, e i Paesi che non intendono condividere le responsabilità dell'accoglienza non dovrebbero essere ammessi ai finanziamenti dell'Unione. Grazie, UV))*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, il nostro augurio è che dal vertice di Bruxelles lei possa tornare con buone notizie per l'Italia. Per quanto riguarda l'immigrazione, gli eventi hanno dimostrato l'inefficacia degli accordi di Dublino, così come l'idea della distribuzione delle quote di migranti. Bisogna continuare a stringere accordi con i Paesi d'origine e con quelli di transito. Dico «bisogna» perché così è stato fatto - anche molto efficacemente - dal Governo Gentiloni Silveri, dall'allora ministro Minniti *in primis.* Bisogna soprattutto lavorare per la costituzione di *hotspot* nel Nord Africa: solo così ci può essere la *governance* di un fenomeno che richiede l'impegno di tutti e su cui l'Italia non può più essere lasciata sola. Francia e Germania si spendano non solo sul tema dell'immigrazione secondaria, ma anche per la gestione della complicata partita dei rimpatri per chi è sprovvisto dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, come richiesto anche dalla Conferenza Stato-Regioni, su iniziativa del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano. Allo stesso modo, ci vuole un'azione corale sulla Libia affinché accetti la costruzione degli *hotspot*. Questi non fanno solo l'interesse europeo ma anche libico, in un'ottica di contrasto alle organizzazioni criminali e del traffico dei migranti. Signor Presidente del Consiglio, le immagini dei bambini separati dai genitori al confine tra Messico e Stati Uniti hanno sconvolto l'opinione pubblica. Per noi ci sono obblighi di carattere umanitario che bisogna sempre rispettare e a cui l'Europa non deve venire meno; per farlo c'è bisogno dell'impegno di tutti. Il vertice di Bruxelles ha altri punti all'ordine del giorno che riguardano la competitività e l'innovazione digitale: non sono temi e obiettivi che intrecciano da vicino le politiche di crescita che il suo Governo intenderà mettere in campo. La guerra sui dazi, la fine delle misure di sostegno della Banca centrale europea, le tensioni internazionali rischiano di rallentare una crescita internazionale nella quale l'Italia non ha brillato per via di una serie di limiti e di ritardi strutturali che risalgono a ben prima della crisi economica. Le raccomandazioni che l'Unione ha inviato a maggio al nostro Paese vanno prese in considerazione, dalla lentezza del nostro ordinamento giudiziario ad un quadro di norme che, in taluni ambiti, è un freno alla competitività e allo sviluppo. Noi dobbiamo rimuovere questi ostacoli per mettere il tessuto imprenditoriale nella possibilità di investire, di assumere, di puntare sull'innovazione di processo e di prodotto. Gli impegni che probabilmente usciranno dal vertice di Bruxelles sulla digitalizzazione, il contrasto all'evasione fiscale, la sicurezza informativa e il commercio ci indicano la strada anche per le riforme verso cui deve andare il Paese. Attendiamo per questo i decreti, più volte annunciati dal Governo. Sono passate già alcune settimane. È giunto il momento di entrare nel merito.

la lettera di intenti per partecipare al progetto intergovernativo di difesa europea. L'Italia quindi è assente all'European intervention iniziative, una forza di intervento rapido promossa dalla Francia ed alla quale appartengono già nove Paesi. Ne cito solo quattro: Germania, Francia, Belgio e Olanda, ai quali aggiungo, quasi incredibilmente, la presenza del Regno Unito, nonostante le scelte antieuropee contenute nella Brexit. Insomma sono presenti tutte le grandi forze militari e l'Italia è assente - lo ripeto - mentre forse sta nascendo una lega di Stati che ambisce a sviluppare una forma di coordinamento rapido e di reattività militare. L'European 12, infatti, si prefigge lo scopo di pianificare congiuntamente gli scenari di crisi internazionale che potrebbero minacciare la sicurezza europea. La difesa europea è una necessità ed è la geopolitica che attribuisce all'Europa una funzione cruciale di baricentro mentre si modificano gli interessi strategici mondiali e le destabilizzazioni a diverse latitudini del mondo e mentre si discute su come fronteggiare le ondate migratorie provenienti dai Paesi africani. L'European 12 ambisce ad un progetto di difesa europea e lo fa nella consapevolezza collettiva di un'antica ambizione strategica rimasta insoddisfatta, ovvero una forza comune europea e una integrazione strutturale delle Forze armate dell'Unione. Attualmente si tratta - è vero - di uno strumento in fase embrionale l'adesione al quale viene descritta in termini flessibili e non vincolanti - cito testualmente - e se questo costituisce un elemento di debolezza, debolezza, rappresenta invece un elemento di forza il numero ristretto dei suoi partecipanti: 12 i Paesi previsti, un numero quindi ridotto rispetto ai 25 della PESCO che lei ha citato, un organismo di cui l'ampiezza ma anche gli interessi geopolitici diversi dei Paesi membri rendono difficile il coordinamento. È per questo che la Francia ha proposto l'European 12 e pur avendo Fratelli d'Italia fortemente criticato gli atteggiamenti, le dichiarazioni e le prese di posizione del presidente Macron sulla questione Aquarius e non solo, più in generale sulla responsabilità europea della questione migratoria, nonostante la nostra posizione, noi giudichiamo grave che l'Italia sia assente, autoescludendosi dalla discussione sul futuro militare dell'Europa e lasciando vuota quella sedia dove discuteranno e si siederanno altri *partner* europei e della NATO. Noi non sappiamo se questo strumento sarà efficace o no ma non lo sa neanche il Governo che ha deciso di non esserci e che non ha ritenuto di dover informare né l'Aula, né il Paese su una scelta così strategica e ci chiediamo anche come si concili tale tale assenza con i nodi fondamentali che l'Italia va a discutere a Bruxelles. Evidentemente mi riferisco a difesa e sicurezza, quella che si vuole rafforzare. E come si farà a parlare di blocco navale, questione che Fratelli d'Italia considera fondamentale e urgente per impedire l'arrivo di navi cariche di immigrazione clandestina? E come potrà ancora l'Italia partecipare e decidere se non si siede ai tavoli? Chiediamo a lei, signor Presidente del Consiglio, se il Governo italiano considera necessario un esercito europeo e se la difesa e la sicurezza europee sono una priorità della nostra politica

oggi un importante commentatore finanziario, parlando del prossimo Consiglio europeo e dell'annesso Euro Summit, affermava, senza esagerare, che si potrebbe dire che si tratterà di un *summit* di portata costituente. Infatti, mai, fino a oggi, il Consiglio europeo aveva avuto all'ordine del giorno due *dossier* di questa importanza: la regolamentazione delle migrazioni e la riforma dell'unione economica e monetaria, nella duplice veste di unione bancaria e misure per l'eurozona. necessitano di una notevole attenzione, soprattutto per l'importanza che noi dobbiamo riporre in fase ascendente, essendo la parte in cui noi partecipiamo, alla formazione del diritto europeo. Dirò di più: su entrambi i punti deve prevalere la consapevolezza, da parte di tutti, che solidarietà e responsabilità... *(Brusio).* PRESIDENTE. Colleghi, il brusio ha superato il limite di guardia e non riusciamo a sentire il collega che parla.

e che si tradurrà in un piano di riforma della zona euro e si concentrerà fondamentalmente su due temi. Analizziamo i due temi. Il primo il ruolo futuro del meccanismo europeo di stabilità. Abbiamo visto che la Commissione ha espresso un giudizio positivo sulla proposta franco-tedesca. Bisogna dire che, per la prima volta in dieci anni, vi è stato uno sforzo congiunto per rafforzare l'integrazione europea. Questo è positivo anche per noi. Creare un bilancio nella zona euro entro il 2021 è una cosa che non possiamo che valutare positivamente, pensando, ad esempio, che la Germania era contraria. Noi sappiamo come questo serva a rafforzare la competitività, rilanciando gli investimenti e come sia stato chiesto con forza dall'Italia negli ultimi quattro anni, in particolare dal Partito Democratico. per il momento, non se ne precisa l'ammontare e - soprattutto - se deve essere inglobato nel bilancio comunitario, oppure no. Ci sono poi diversi altri punti che, invece, non possono essere accolti, *in primis* la condizionalità cui sarebbe sottoposto l'intervento dell'ESM se si trasformasse in Fondo monetario europeo. Agirebbe, nei casi di difficoltà di un Paese, solo previa ristrutturazione del debito e ciò finirebbe per dare un potere non indifferente a Francia e Germania sulle decisioni del Meno peggio il potenziale accordo perché il meccanismo europeo di stabilità dell'ESM diventi il paracadute del Fondo di risoluzione unico, anche se la dotazione data effettivamente viene ritenuta ancora troppo bassa, nonostante, anche su questo, la Germania non fosse d'accordo. Il secondo punto, come è emerso anche in altri interventi, penso rappresenti il vero e proprio problema: il completamento dell'unione bancaria. Dopo il primo pilastro - il meccanismo unico di vigilanza - e il secondo pilastro - il meccanismo di risoluzione unico, che è partito dal 1° gennaio 2016 - non possiamo accettare che non si arrivi alla realizzazione, nel più breve tempo possibile, del terzo pilastro. Mi riferisco al Fondo di risoluzione unico, che è stato solo abbozzato attraverso un percorso che è di una complessità eccessiva. La prima fase è quella del meccanismo del cofinanziamento, la seconda fase è quella del meccanismo della coassicurazione e solo nella terza fase si arriverebbe allo schema europeo di garanzia dei depositi bancari (EDIS). Questo non va assolutamente bene. Purtroppo nella riunione dei 27 dell'Eurogruppo del 21 giugno scorso è stata ribadita la necessità di un approccio graduale e penso che questa dichiarazione sia stata fortemente condizionata dal vertice franco-tedesco di che ha introdotto un principio che porta ad una sequenza della riduzione dei rischi e della condivisione degli stessi. Ebbene, questo è ancora un aspetto secondario ma molto grave, se lo poniamo in relazione all'obiettivo che vuole essere introdotto di ridurre

che è riuscita a creare le condizioni per passare in un anno, dal 2017, da uno stato di 230 miliardi lordi a uno di 186. In questo ci sta la valutazione di quello che di sequenza, che deve tenere nella stessa considerazione sia la riduzione dei rischi, sia la condivisione. Se non si fa questo, il processo finisce per essere un processo monco, ma soprattutto non si dice

dalle banche francesi e il 30 per cento dalle banche tedesche. Va bene allora rafforzare l'eurozona, va bene non danneggiare gli interessi nazionali, ma penso che dobbiamo porci come obiettivo quello di creare le condizioni perché non si presenti il pericolo di titoli liquidi (gli L2 a cui a cui faceva riferimento la senatrice Bottici). Quanto prima il senatore Parrini diceva che non abbiamo visto cambiamenti tangibili, devo dire che invece un cambiamento tangibile l'ho visto perché due anni fa non lei, ma il MoVimento 5 Stelle queste cose non le avrebbe mai dette. In conclusione vorrei una domanda al nostro Presidente del Consiglio. Io non penso che il Governo italiano sia disposto ad accettare questo pericolo, ma il rischio è di doverlo fare per due motivi: o a causa della debolezza dei conti o a causa, a leggere i giornali dell'altro giorno, della necessità di ottenere concessioni sul *deficit* per poter realizzare promesse elettorali in una visione di scarsissimo respiro per il bene del Paese. Ebbene, Presidente, facendole un'apertura di credito, sono convinto che lei si opporrà - utilizzando le parole che ha pronunciato prima - con la forza e la consapevolezza di un Governo che in Europa parla con una voce sola, ferma e risoluta, farà in modo che questo non avvenga, anche se - da quello che ho visto per ora - ho qualche ragionevole dubbio che ciò possa avvenire.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Italia ha finalmente assunto un ruolo propositivo e attivo in Europa. L'Italia, guidata da un Governo che si è insediato da pochi giorni, ha finalmente alzato la voce. È stato necessario farlo, per invertire la rotta dopo anni di politiche servili verso gli Stati esteri, in particolare verso il cosiddetto asse franco-tedesco. L'obiettivo dichiarato della proposta italiana è colmare le evidenti lacune delle politiche finora attuate nell'ambito dell'Unione europea in materia di immigrazione e asilo, politiche che hanno, di fatto, portato alla situazione di grave emergenza che stiamo subendo: una emergenza strutturale. Secondo i dati resi noti dal Ministero dell'interno a cura del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, dal 2013 al 2017 su oltre 600.000 arrivi registrati solo via mare in Italia, le domande di protezione internazionale complessivamente presentate sono in numero inferiore (429.195), e di quelle esaminate oltre la metà hanno ricevuto un diniego dalle Commissioni territoriali. Sempre secondo gli stessi dati, dal 2013 al 2017 la media delle domande di protezione internazionale accolte a cui è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato è stata del 7,2 per cento, media confermata anche per le domande esaminate quest'anno dalle Commissioni territoriali. I dati non sono suscettibili di interpretazioni: l'Italia è diventata la meta privilegiata di un flusso migratorio composto principalmente da migranti economici, e solo in una minima parte da persone in fuga dalle guerre e bisognose di aiuto. Questo flusso è stato gestito, negli ultimi anni, in maniera fallimentare. L'Unione europea ha scaricato sull'Italia sia il peso della difesa dei confini dai clandestini (confini che sono sì italiani, ma anche europei), sia l'onere di accogliere chi ha realmente bisogno di un Paese dove rifugiarsi perché perseguitato politicamente. ad esempio, al programma di ricollocamento dei richiedenti asilo proposto dalla Commissione europea e adottato con due decisioni del Consiglio UE nel settembre 2015. Esso prevedeva in due anni, ossia entro settembre 2017, il ricollocamento di 160.000 richiedenti asilo da Italia e Grecia negli altri Paesi europei in base a un sistema di quote. Secondo i dati disponibili ad oggi risultano ricollocati dall'Italia in altri stati dell'Unione europea solo 12.722 richiedenti asilo sui 34.953 previsti. Un terzo di quello che dovevamo aver ricollocato. E molto altro ci sarebbe da dire, soprattutto su chi recentemente non ha perso occasione per farci la morale. Quanto meno abbiano il buon senso di tacere! Il Trattato di Dublino, nato prima come Convenzione tra Stati e poi divenuto Regolamento in un'epoca diversa rispetto a quella odierna, non è più adeguato a far fronte alle attuali esigenze. Parlare della posizione favorevole che la Lega espresse al tempo nei confronti del trattato, quando la situazione geopolitica e sociale era totalmente differente, è parlare a sproposito. Infatti, il principio del Paese di primo approdo era stato concepito come criterio responsabilizzante per per i Paesi europei, affinché presidiassero adeguatamente i loro confini. Oggi, invece, i confini ce li avete fatti abolire. L'esiguità dei flussi migratori lo esigeva. Ma ora le forti pressioni sui nostri confini marittimi (e su quelli degli altri Paesi mediterranei) impongono una completa revisione di tale sistema: revisione che impone il rafforzamento e il presidio dei confini comuni. Molti esponenti dell'opposizione rivendicano di aver portato avanti negli anni passati una linea simile a quella presentata dal Governo. Dunque, mi permetto di concludere con un concetto molto semplice: i buoni propositi diventano azioni concrete soltanto se vengono realizzati. Ed è molto più probabile che il problema strutturale del flusso migratorio

signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, il Consiglio europeo ha tra gli altri temi in esame quello del bilancio pluriennale dell'Unione europea. Si tratta di una programmazione che va dal 2021 al 2027 e che pure verrà marginalmente affrontata in un'agenda ricca di altri punti. 1.135 miliardi di euro di stanziamenti pari all'1,11 per cento del reddito nazionale lordo dell'Unione europea a 27 membri nei sette anni. Ed è utile ricordare che l'Italia è uno dei cosiddetti contributori netti del bilancio europeo. Questo significa che versa alle casse di Bruxelles più di quanto poi riceva attraverso i vari fondi comunitari per le Regioni, la ricerca, lo sviluppo, i migranti e tutte le altre politiche comunitarie. Questo deve essere sempre un particolare che va rammentato ai *partner* europei, soprattutto quelli che in questi anni hanno beneficiato dell'adesione dell'Italia al progetto europeo. Nel 2016, ultimo anno per cui abbiamo i dati, l'Italia ha versato nelle casse di Bruxelles 13,393 miliardi di euro. Nel 2015 erano stati 14,691 miliardi; nel 2014 14,594 miliardi e nel 2013 - cifra *record* - di 15,748 miliardi. Per quanto riguarda i miliardi che l'Italia riceve a sua volta dall'Europa, la media si aggira sugli 11,5 miliardi. Nel 2016 sono stati 11,592 miliardi;

Il «saldo» è stato, insomma, sempre ed effettivamente negativo in questi anni rispettivamente di 1,8; 2,35; 3,9 e 3,2 miliardi, per una media di 2,8 miliardi. Secondo la Relazione che la Corte dei conti ha riservato ai «Rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi comunitari» nel periodo 2010-2016 il contributo complessivo netto italiano all'Europa è stato il quarto, dopo Germania, Regno Unito e Francia, mentre solo una parte delle risorse ricevute dal nostro Paese è arrivata effettivamente sui nostri territori. Ho fatto queste premesse con un po' di numeri proprio per dare un ritratto del rapporto che vincola l'Italia all'Europa, dalla quale riceviamo soprattutto, ogni anno, centinaia di disposizioni da recepire nel nostro ordinamento attraverso apposite leggi o magari inserite nei meandri dei vari decreti. Nell'ambito della nuova programmazione 2021-2027 noi di Forza Italia temiamo che l'Italia possa subire una nuova forte penalizzazione, soprattutto in conseguenza dei tagli previsti dall'Unione ai fondi per l'agricoltura e al Fondo di coesione. Queste riduzioni, in attesa di capirne esattamente l'entità, non possono certo essere compensate dai maggiori contributi destinati all'immigrazione, di cui pure si parla, che non andrebbero a coprire che una piccola parte di quei maggiori oneri. Proprio sui temi importanti come le risorse per l'agricoltura e la pesca e i fondi di coesione bisognerà agire per tutelare l'interesse nazionale al tavolo del Consiglio: Consiglio: alcune stime parlano infatti di tagli alle Regioni dal Fondo di coesione in termini reali che sfioreranno il 10 per cento. Vi è poi l'allarme relativo a uno dei criteri di distribuzione delle somme - e cioè il PIL *pro capite* delle Regioni che potrebbe penalizzare sensibilmente alcune Regioni a discapito di altre che, appunto, hanno un PIL sotto il 75 per cento della media europea. Anche per i tagli ai fondi per l'agricoltura la situazione appare ben più critica di quanto non dicano i dati diffusi dalla Commissione. Il taglio per gli agricoltori del *made in Italy* si potrebbe tradurre in circa 20 miliardi complessivi per il settore nel periodo della nuova programmazione. A pagare le conseguenze di questa Europa che cambia marcia saranno le politiche agricole e quelle di coesione e, di conseguenza, potrebbero essere sensibilmente ridotti i fondi destinati agli enti territoriali, alle piccole e medie imprese e ai giovani. In questo ambito bisognerà stare attenti che anche la montagna, le zone di confine e le loro peculiari problematiche non abbiano a subire ulteriori penalizzazioni. In alcune Regioni si devono affrontare i più svariati problemi, come quelli dell'agricoltura di montagna o la questione dei grandi carnivori. A tal proposito sottolineo che la Convenzione delle Alpi, trattato territoriale internazionale tra i Paesi alpini e l'Unione europea, rappresenta la volontà di equilibrare le necessità e le esigenze dell'uomo con lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente naturale. Ci sono poi i più recenti progetti Life WolfAlps e Life Ursus, promossi dall'Unione europea, atti a salvaguardare due specie protette *ursus *ursus arctos* e *canis lupus*, che purtroppo negli ultimi periodi stanno minacciando i nostri alpeggi che sono una grande risorsa fondamentale per la cura del territorio montano con un importante risvolto anche nel settore turistico di montagna. Occuparsi dei grandi carnivori significa occuparsi, non solamente di specie animali, ma anche di persone, specialmente di agricoltori e di pastori, che sono parti interessate ad affrontare un rischio reale proprio per la presenza di queste specie (grandi carnivori). Bisogna intervenire per tutelare nell'insieme l'uomo, la natura La Politica Agricola Comune rimane un modello basato su competitività e innovazione. Noi, al contrario, dobbiamo puntare su un modello che prediliga la qualità, concetto che spesso contrasta con la quantità. Dobbiamo ascoltare le ragioni e le preoccupazioni dei nostri territori e dei nostri agricoltori, che magari ci evidenziano le loro angosce per un accordo come il CETA e per le ripercussione che potrebbe avere sulle nostre produzioni e sulla qualità dei prodotti, che finiscono sulla tavola dei consumatori. Inoltre va rammentato che ci sono soprattutto territori che vanno fieri delle proprie radici storiche, culturali e di appartenenza a minoranze linguistiche, come quella ladina, di cui mi onoro di far parte e che mi onoro di rappresentare nel mio territorio. Infatti in Europa si contano numerose minoranze linguistiche, riconosciute e tutelate dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie...

Insomma, presidente Conte, dobbiamo chiedere un'Europa che affronti la complessità dei nostri territori e che rappresenti appieno la loro ricchezza culturale e linguistica e la larga varietà delle nostre genti e della nostra produzione.

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, intervengo in questo importante dibattito portando all'attenzione due temi, quello dell'insularità e quello delle infrastrutture di ricerca, che ben si inseriscono all'interno della riflessione che ha fatto nel suo discorso introduttivo a proposito dell'identità dell'Europa e della coesione interna. A proposito di cultura, un gruppo di scienziati italiani, in stretto contatto con colleghi europei e internazionali, ha messo a punto l'interferometro Virgo, per lo studio e la misurazione delle onde gravitazionali, capaci di svelare quel 96 per cento del nostro universo ancora invisibile. Si tratta di una nuova rivoluzione scientifica, di importanza pari a quella avviata da Galileo più di trecento anni fa. Il telescopio Einstein è un osservatorio di terza generazione, capace di raggiungere una sensibilità tale da esplorare un volume del cosmo 1.000 volte più grande di quello che potranno sondare i rivelatori interferometrici attuali. 580 scienziati europei hanno sottoscritto una lettera di intenti per la realizzazione del primo Centro europeo per la misurazione delle onde gravitazionali. È essenziale, signor Presidente, che il progetto rientri ufficialmente nella *road map* European strategy forum on research infrastructures (ESFRI), poiché nell'agosto del 2019 sarà scelto quello migliore e il progetto italiano ha già individuato come localizzazione ideale un sito nella Sardegna centrale, a Lula, in prossimità della miniera dismessa di Sos Enattos, assolutamente quieto, sia dal punto di vista delle attività umane

poiché la candidatura di questa importantissima infrastruttura di ricerca viene effettuata dagli enti proponenti (università, Istituto nazionale di fisica nucleare, Istituto nazionale di astrofisica), col supporto di almeno tre Governi, di cui uno si proponga come guida e capofila. I nostri competitori sono due: da una parte ci sono Olanda, Germania e Belgio, che hanno individuato un sito in una striscia di terra confinante tra tre Nazioni e dall'altra c'è il progetto ungherese. Le caratteristiche del progetto italiano sono però, a detta degli esperti, di gran lunga migliori sotto ogni punto di vista. Ciononostante, signor Presidente, non vorremmo assistere ancora una volta impotenti a logiche lobbistiche, che poco hanno a che fare con la qualità dell'iniziativa e che finiscono solo col mortificare la comunità scientifica italiana. Creare centri di ricerca di questo livello significa, signor Presidente del Consiglio, invertire la triste realtà della fuga di cervelli, offrendo invece concrete opportunità di lavoro ai ricercatori e al personale tecnico specializzato. Realizzare queste infrastrutture in un'area tra l'altro fortemente depressa e a forte rischio di spopolamento - mi sia consentito dirlo da sardo - è una formidabile occasione di crescita cui dovranno seguire necessariamente altri interventi per colmare le distanze derivanti dall'isolamento. *(Commenti dal Gruppo PD).* Proprio sul tema dell'insularità vorrei richiamare la sua attenzione, visto che il bando europeo per garantire la continuità territoriale la continuità territoriale rischia di lasciare la Sardegna priva di collegamenti aerei a partire dal mese di ottobre, con grave danno per l'economia. Come è noto, le politiche di concorrenza dell'UE garantiscono che le imprese competano in modo leale e in condizioni di parità nel mercato interno europeo; d'altro canto, la stessa Unione europea riconosce in vari trattati e documenti la situazione di svantaggio oggettivo derivante dalla condizione di insularità, sotto il profilo del *surplus* dei costi dei trasporti, dei costi energetici, nonché dell'accesso al mercato, in particolare delle piccole e medie imprese. Noi non vogliamo assistenza, ma giustizia. Io le chiedo di inserire questi due punti: il primo riguarda la ricerca scientifica a livello europeo il secondo punta a risolvere il problema della insularità, a dare effettività ai documenti espressi dalla Unione europea. Signor Presidente del Consiglio, le auguro un buon lavoro nella certezza che ella saprà tutelare al meglio la posizione italiana nel prossimo Consiglio europeo.

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, nei pochi minuti a mia disposizione mi soffermerò solo sulla parte del suo intervento che riguarda la questione migratoria, un punto chiave della discussione odierna

dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e approvato in quella sede. C'è bisogno, infatti, di un sistema di regole chiare per il riparto nazionale dei richiedenti asilo che giungono in Italia, non solo via mare ma anche via terra, da altri Paesi europei. Per questi migranti, a differenza di quelli che giungono via mare, non vi è infatti un criterio di attribuzione tra le Regioni e credo che questo debba essere oggetto di attente valutazioni prima e in vista del vertice di Bruxelles. Una seconda considerazione la questione migratoria ha un particolare impatto sulla Provincia autonoma di Bolzano, con specifico riferimento alla frontiera del Brennero. Come è noto, l'Austria, di fronte al flusso migratorio, ha minacciato la chiusura del Brennero. Tale chiusura rappresenterebbe un grave passo indietro e inciderebbe negativamente non solo sulle buone relazioni tra l'Italia e l'Austria, ma anche sulla libera circolazione dei cittadini, sul turismo, sugli scambi commerciali e quindi sull'intera economia. Su questi punti ci aspettiamo un confronto costruttivo a livello europeo che porti a una soluzione comune e condivisa. L'augurio è quindi che possano giungere finalmente buone notizie. Andare oltre l'accordo di Dublino è fondamentale, come lo è anche il fatto che ogni Paese faccia la sua parte.

per la correttezza istituzionale che ha mostrato nel voler seguire l'intero dibattito, correttezza istituzionale che non è una materia primaria e in grande spolvero in questo periodo nel nostro Paese. Non sono una catastrofista di carattere e neanche una pessimista; sono testarda e un po' cocciuta. Eppure ho seguito la preparazione di questo vertice, come di quello di domenica scorsa, con enorme preoccupazione. Non solo per il linguaggio: mai ho assistito a un livello di insulti di questo tono tra Capi di Stato o Ministri dell'Unione europea. E se così vi trattate, come pensate che si deve trattare la gente al bar? Ma non sta a voi dare l'esempio di un po' di misura, nell'usare le parole giuste, parole che

L'ho seguita con grande preoccupazione, perché vedo avvicinarsi un vertice che sarà un passo in avanti - temo - nello sgretolamento dell'Unione europea intergovernativa, che è sempre quella che non funziona. Mentre funzionano le politiche comunitarie - su cui uno può dissentire nel merito e volerne altre le politiche intergovernative, quelle previste dai trattati e quelle che vi siete autoattribuite, sono un disastro, vertice dopo vertice.

Ma vi pare davvero che, se noi insistiamo «in prima i maltesi», «prima gli ungheresi», «prima i francesi» - ovviamente - e «prima gli italiani», andremo mai da qualche parte? Forse, se provassimo a guardarci in faccia e a dirci «prima le persone», nella legalità e nel rispetto delle convenzioni, nel rispetto dei diritti e dei doveri,

una politica comune sull'immigrazione sono sempre stati gli Stati membri, salvo implorarla quando tocca a qualcuno di loro. Chi non ha mai voluto la protezione europea delle frontiere esterne sono sempre stati gli Stati membri, salvo poi invocarla quando conviene e di volta in volta. Penso, signor Presidente, che nessuno più di noi, più di me (e da tempi non sospetti), quanto le regole europee in materia di immigrazione siano, da un lato, insufficienti e, dall'altro, superate dai cambiamenti strutturali cui assistiamo da tempo. Ricorderò sempre il vertice di Tampere del quando l'Italia (il presidente Napolitano, insieme ad altri) chiese una politica europea dell'immigrazione. Il commissario Vitorino la propose e fu cacciato a furor di Stati membri. Quindi credo che mettere riparo e trovare canali legali di ingresso sia il tema da affrontare, insieme con la

Penso che si stia arrivando veramente allo sgretolamento dell'Europa intergovernativa, che si porterà dietro anche il fallimento dell'Europa comunitaria. Mi auguro di sbagliare e spero che non sia così. Posso anche dire che nel documento complesso che ho presentato, e che i suoi uffici, signor

e vedrà giovedì e venerdì, che con gli *slogan* non si va da nessuna parte. Quella che stiamo affrontando era, semmai, una crisi umanitaria, che invece è diventata, per ragioni di consenso, una crisi politica,

allo stadio, non è il due più uno. Io capisco e lei si troverà a dover negoziare, e spero lo faccia, perché così si fa all'interno dell'Unione europea Un po' di calma e ho chiuso. Impeti e furori di linguaggio, di che parla di pacchia, di crociere, di centri di prim'ordine in Libia, avendone visitato uno che non è ancora neanche in funzione. Oppure chi mi parla di retorica delle torture: guardate qualche fotografia e pensate se foste voi o se fosse qualcuno della vostra famiglia! Infine, calmi un attimo: lei è il Presidente del Consiglio, ci sono Ministri un po' straripanti, diciamo così, quelli che magari non hanno tempo di andare a convincere Orban e i suoi amici, ma hanno tempo ogni giorno

Lei è il Presidente del Consiglio, l'articolo 92 della Costituzione è chiaro: la divisione delle competenze è uno dei pilastri fondamentali e portanti del nostro Viva Europa, e lo dico. Lei sa che l'alternativa non c'è; l'alternativa è: 28 Paesi allo sbando, ognuno per conto suo, quando dall'altra parte avete la Cina, Trump

E non è il caso di chi urla più forte; è il caso di chi è più credibile.

il tema della migrazione è sicuramente, come si è visto anche dagli interventi di coloro che mi hanno preceduto, un tema centrale per quanto riguarderà la posizione del nostro Paese al prossimo Consiglio europeo.

su determinati aspetti del tema della migrazione. Abbiamo apprezzato la chiusura dei porti, l'aver avuto il coraggio di rispondere in modo diverso al buonismo che ha caratterizzato la politica degli ultimi anni della sinistra italiana. Abbiamo apprezzato questo, come abbiamo apprezzato il fatto che abbiate ammonito le navi delle ONG, di quei trafficanti di esseri umani che il buonismo delle sinistre ha favorito. *(Applausi dal Gruppo

Abbiamo apprezzato l'intento che lei oggi ha dichiarato, signor Presidente del Consiglio, di attivare degli accordi con i Paesi del Nord Africa, con i Governi della Libia.

Signor Presidente del Consiglio, voglia però accettare questo invito ad avere maggior coraggio nel prossimo vertice del 28 e 29 giugno; maggior coraggio, perché l'Italia deve far valere il proprio *status* e il proprio diritto. Non possiamo e non vogliamo diventare il campo profughi dell'Europa. Qualcuno vicino al presidente Macron Macron ha definito «vomitevole» la posizione del Governo italiano; io rispondo che vomitevole è la posizione dei francesi e di coloro che in questa fase

Il concetto è che serve un presidio delle frontiere, serve subito un blocco navale. E non mi si dica da sinistra che non è possibile, perché nel 1997 fu Prodi ad attuarlo in Albania. L'Europa tutta unita, quindi, si attivi per un blocco navale, per un presidio delle frontiere. Ecco perché - concludo, Presidente - noi siamo a favore dei Paesi del Fratelli d'Italia è coerente con chi le proprie frontiere le ha difese sui Balcani, quindi non può accettare di vedersi redistribuire quei profughi che qualcun altro, collaborando con le ONG, aveva accolto. per la quale Fratelli d'Italia, con forza, chiede a questo Governo di allinearsi con chi difende le frontiere, cioè con Visegrád, con chi difende la nostra civiltà, la nostra religione, la nostra cultura e la nostra economia. *(Applausi

intende svolgere nel processo d'integrazione europeo. Come ricordava la senatrice Bonino, le attuali tensioni, infatti, rischiano di minare persino il più flessibile degli scenari immaginati appena qualche tempo fa dalla Commissione europea nel suo Libro bianco sul futuro dell'Europa. Tensioni interne, cui si aggiungono sfide decisive nel panorama geopolitico internazionale in rapida evoluzione, e che riguardano il rischio stesso di isolamento politico dell'Unione europea, tra neoprotezionismi commerciali e neosovranismi politici. Per questo noi riteniamo sia necessario accelerare sul terreno dell'integrazione, ma anche sul terreno dell'allargamento, in un'Europa che rischia di dividersi tra un nuovo Est e un nuovo Ovest, tra populismi e neonazionalismi dopo oltre sessant'anni di pace e di sviluppo. Siamo noi i primi a invocare un passo in avanti dell'Europa, di un' altra Europa, quella dei popoli, che recuperi il sogno di Ventotene, le ragioni ideali di quel progetto e che rimetta al centro le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini. Per recuperare un'autentica legittimazione democratica riteniamo pertanto necessario, accanto alla modifica della *governance* istituzionale, spingere l'acceleratore del pilastro sociale, di cui lei non ha fatto cenno, sottoscritto anche dall'Italia al vertice di Goteborg nel novembre scorso, e affrontare le tante storture e disuguaglianze generate dalla crisi che abbiamo appena lasciato alle spalle. E allora, accanto al tema dell'unione bancaria, del Fondo monetario europeo e di un ministro delle finanze per la zona euro, vorremmo che si chiedesse che i principi di tutela sociale divenissero obblighi di derivazione europea; che i diritti sociali vengano quindi integrati nella procedura stessa del semestre europeo, anche in relazione alla formulazione delle raccomandazioni specifiche per il Paese, per una crescita che sia effettivamente inclusiva e cioè capace di generare occupazione. Siamo d'accordo, anche prevedendo sussidi europei contro la disoccupazione e a sostegno del reinserimento lavorativo. Maggiore protezione e maggiore sicurezza di fronte a fenomeni che solo a livello europeo che solo a livello europeo possono trovare la dimensione per una risposta efficace, verso la creazione di uno spazio unico interno di libertà, sicurezza e giustizia, ma a cui corrisponda necessariamente - e anche noi siamo d'accordo - un controllo più forte e maggiormente integrato della frontiera esterna europea, verso una comune difesa europea. È quello che noi abbiamo fatto con le operazioni coordinate dalla Guardia costiera europea per richiamare a responsabilità i diversi Paesi membri dell'Unione sul tema della gestione dei flussi migratori. È sulla conciliazione e non sulla contrapposizione di sicurezza e solidarietà che è necessario dare completa attuazione al Trattato di Lisbona verso una comune politica di immigrazione e di asilo, certo superando definitivamente il principio della competenza del Paese di primo ingresso di una Convenzione, quella di Dublino, sottoscritta dal Governo di centrodestra nel 2003 e che noi, già dal 2015, abbiamo chiesto di superare. La Convenzione di Dublino, infatti, combinata con gli effetti della vostra legge Bossi-Fini, costringe costringe il nostro Paese a una condizione di difficoltà nella gestione dei flussi perché, di fatto, trasforma tutti i migranti in ingresso in richiedenti asilo,

dove siamo riusciti a rimpatriare 25.000 migranti con il rimpatrio assistito e volontario. Voi non avete fermato gli arrivi e gli sbarchi. Noi abbiamo fermato, colpendo con l'economia,

se stare accanto ai Paesi di Visegrád, con l'Ungheria di Orban, oppure stare con i Paesi che vogliono un'Europa più forte e una difesa comune. In questo momento, dopo la Brexit, forze della disgregazione sono al lavoro per minare l'edificio europeo. A noi ci troverete sempre sul fronte opposto. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori del Governo, vi attende un altro importante appuntamento dove lei, presidente Conte, è chiamato a consolidare la nostra posizione sui temi che prima ha già ampiamente citato e anche sul nostro ruolo di fondatori dell'Europa; fondatori, ma non più disposti a diventarne vittime. L'Europa è, infatti, bloccata da tempo, come afflitta da una paralisi politica identitaria, presidente Bonino, perché vinse l'idea della Francia, ancora una volta, anche quella volta: l'Europa delle Nazioni e non delle politiche. Le Nazioni europee tendono a non distruggere quanto costruito, aggiustando sul piano politico i difetti tecnici del modello, senza mai però riuscire senza mai però riuscire a ripararli, soprattutto sul modello monetario, croce e delizia di questa Europa. La convergenza - l'unica cosa possibile - si realizza nel non distruggere,

che abbiamo ascoltato anche negli interventi che mi hanno preceduto: in Italia impegnati a combattere l'elusione e l'evasione fiscale - come lei ha ricordato, presidente - inondando i nostri cittadini di cartelle di Equitalia, pazze o non pazze, e in Europa a consentire il vile *dumping* fiscale di Lussemburgo e Olanda in nome dell'unione fiscale. In Italia a svendere le banche nel territorio, previa azione mirata delle tante vigilanze che il presidente Marino prima ha ricordato;

minori e di qualità certamente diversa perché legata all'economia reale del territorio, dovessero sparire magicamente in dodici mesi, giusto per svenderle meglio a qualcuno di particolarmente interessato. Altro che unione bancaria, vi ha ricordato prima il collega Bagnai. Lei ha già detto benissimo, presidente Conte, che è forte la nostra contrarietà a un Fondo monetario europeo, che somigli magari ad altri Fondi monetari che hanno accompagnato le sventure di tanti Paesi nel mondo, che esautori gli Stati membri del perseguimento di politiche economiche efficaci. Per l'Italia forse si riapre la possibilità di recuperare, grazie anche a questo, un ruolo paritario nella *governance* europea e di spingere l'Europa - quella vera - verso una rinnovata alleanza con i suoi cittadini e, per esempio, con gli Stati Uniti d'America nel nuovo quadro geopolitico che - i tempi ci hanno dimostrato - cambia. È forse per questo che si ripetono le provocazioni francesi

consentire che le provocazioni e gli insulti al Governo italiano facciano dimenticare quegli interessi contrastanti della Francia contro l'Italia sulla questione migratoria scatenata dalle rinnovate mire economiche ed espansionistiche sull'Africa, a cominciare dai fatti accaduti in Libia, o la campagna campagna francese sulle aziende italiane, presidente Conte. Mi riferisco a quelle acquisizioni "magiche" avvenute nel nostro Paese negli ultimi dieci anni: 52 miliardi di euro di valore italiano, di aziende tutte italiane trasferite magicamente in Francia. Al contrario, solo 2,5 miliardi di euro di acquisizioni da parte delle aziende italiane verso le aziende francesi: 52 miliardi contro 2,5 miliardi, che somigliano tanto a quei 640 immigrati contro i 650.000 che questo Paese ha dovuto accogliere

andate in quel Consiglio portando la voce di tutti gli italiani che vogliono essere europei, ma che non vogliono morire d'Europa.

presidente Conte, il Consiglio europeo dei prossimi giorni è sicuramente un *summit* decisivo per il futuro dell'Unione, ma è anche il primo, vero, banco di prova del Governo e delle sue capacità diplomatiche. In questo delicato contesto non si parlerà solo delle politiche di gestione dell'immigrazione, ma anche di come riformare la *governance* economica dell'eurozona, delineandone le nuove regole di funzionamento per i prossimi decenni. Per quanto riguarda l'emergenza immigrazione, Forza Italia da anni sostiene la necessità di individuare con gli Stati membri dell'Unione soluzioni comuni per fronteggiare il problema. Fino ad ora, le misure adottate si sono rivelate insufficienti ed è evidente, quindi, la necessità di cambiare rotta. Certo, comprendiamo che non esistono soluzioni semplici al problema complesso dell'immigrazione, ma riteniamo che l'Europa tutta, e non solo una sua parte, debba farsene carico; non certo sigillando i propri confini o alzando muri e barriere - rinnegando così la sua stessa essenza - ma lavorando con la consapevolezza che è giunto il momento di iniziare a parlare con una sola voce e di essere un'entità unica, anche se plurale. Le nostre capacità di accoglienza non sono illimitate; riteniamo di poter accogliere solo chi possiamo integrare, perché crediamo sia giusto offrire una vita dignitosa, e non un calvario fatto di umiliazioni e sfruttamento, a chi viene nel nostro Paese. Chi giunge in Italia giunge in Europa, per questo abbiamo sempre sostenuto la necessità di superare il Regolamento di Dublino e il criterio del primo Paese di sbarco. Per la cronaca, lo dico ai colleghi dell'Aula, l'attuale versione del Regolamento di Dublino è stata sottoscritta dal Governo italiano nel 2013, quando Presidente del Consiglio era Enrico Letta del PD. Quando il Governo Berlusconi lo sottoscrisse per la prima volta non c'erano ancora state le primavere arabe e la destituzione del regime di Gheddafi, su cui noi eravamo fermamente contrari. *(Applausi Giusto, quindi, rivendicare una maggiore collaborazione da parte dei Paesi dell'Unione facendo leva sulla necessaria e non più rinviabile dimostrazione da parte di tutti di un maggiore spirito solidaristico. Gli oneri dell'accoglienza non possono più ricadere solo sul Paese di primo sbarco e occorre un meccanismo automatico di redistribuzione dei migranti tra tutti i Paesi dell'Unione per salvaguardare i diritti di chi arriva ed evitare problemi di sovraffollamento e inevitabili tensioni sociali. Occorre lavorare per intensificare le relazioni diplomatiche, gli accordi tra Unione europea e Paesi terzi da cui provengono o transitano i flussi migratori. Bisogna aprire centri di identificazione in questi Paesi e far arrivare in modo sicuro in Europa solo chi ne ha diritto perché fugge da guerre o da persecuzioni. Il drammatico traffico degli esseri umani e il successivo *business* dell'accoglienza devono avere fine. Tra il 2014 e 2017 hanno perso la vita nel Mediterraneo almeno 13.000 persone e l'Unione europea non può più permettere questa carneficina. Seguendo l'esempio dell'accordo con la Turchia che ha chiuso la rotta balcanica, l'Unione europea deve investire almeno sei miliardi di euro per chiudere le rotte del Mediterraneo e seguendo l'esempio della cooperazione tra l'Unione europea e il Niger, dobbiamo cooperare di più con Paesi di transito come Mauritania, Mali, Tunisia, Marocco e Algeria. Serve predisporre, inoltre, un grande piano Marshall a sostegno dei Paesi africani. Abbiamo sempre sostenuto, infatti, la necessità di attivare un piano di aiuti a favore dell'Africa. Da tempo Forza Italia, con il nostro Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ribadisce l'importanza di inserire nel prossimo bilancio europeo aiuti strategici a favore di queste popolazioni che possano metterle nelle condizioni di avere una economia autosufficiente puntando su agricoltura, piccola industria manifatturiera e trasferimento di tecnologie moderne. Ciò detto, presidente Conte, se da una parte crediamo sia sacrosanto rivendicare una maggiore collaborazione e solidarietà da parte dei Paesi membri dell'Unione europea, dall'altra suggeriamo attenzione e minore disinvoltura nell'utilizzo di toni incendiari; incendiari; attenzione all'uso della retorica fine a se stessa, attenzione al continuo ricorso a prove muscolari con l'Europa che rischiano di portarci a un nulla di fatto o peggio di rivelarsi un *boomerang* per il nostro Paese, condannandoci all'isolamento. Siamo contrari alla logica della campagna elettorale permanente. Ciò che adesso deve prevalere è la concretezza e il buon senso. Fare la voce grossa finora non ha portato ad alcun risultato concreto. Non basta chiudere i nostri porti alle ONG. Gli arrivi in Italia continuano ancora perché queste organizzazioni si sono fatte furbe: prendono il clandestino, lo depositano su una nave mercantile e lo fanno comunque arrivare a destinazione. La lotta agli scafisti deve proseguire e non si deve limitare alla chiusura dei porti alle ONG perché alcune di queste organizzazioni continuano ad aiutare gli scafisti che speculano sulla disperazione del continente africano. Governare, Presidente, non vuol dire guadagnarsi qualche titolone sui quotidiani ma dare delle risposte concrete ai cittadini portando a casa risultati di lungo termine. La questione immigrazione è un problema epocale e globale. Non possiamo limitarci a subirlo ma dobbiamo affrontarlo con pragmatismo, evitando di trasformare il confronto dialettico in scontro ideologico, tenendo conto che tutti i partiti politici, da sinistra a destra, non possono non ritenere l'argomento centrale per il futuro del nostro Paese e dei nostri figli. Alla propaganda continua che fa leva sul risentimento popolare, ci auguriamo quindi subentri un impegno serio del Governo nei confronti delle aspettative dei cittadini. Vede, Presidente, un segnale concreto in tal senso il suo Governo potrebbe darlo subito abolendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, un *unicum* nell'Unione europea voluto dalla sinistra che non trova applicazione in nessun altro Paese e che consente ai migranti economici di rimanere in Italia. Al tavolo del Consiglio europeo si discuterà anche delle proposte della Commissione europea per il bilancio 2021-2027. Bruxelles propone dei tagli ad agricoltura, pesca e fondi per la politica di coesione, cioè quelli destinati alle aree più depresse del nostro Paese, *in primis*, naturalmente, quelle del Sud. Se queste proposte si concretizzassero sarebbe una iattura per tutto il nostro Mezzogiorno. Inutile ricordarle, infatti, Presidente, che sarebbe impensabile apportare dei tagli in settori che garantiscono lavoro a moltissimi cittadini del Sud. Ci sono Regioni meridionali che fondano l'80 per cento della loro economia su agricoltura e pesca. Dobbiamo difendere, incentivare e proteggere il lavoro, anziché pensare a misure assistenzialistiche. *(Applausi dal Gruppo non restare a casa ad aspettare i sussidi che lo Stato concede loro. Dobbiamo fare in modo che il Sud Italia possa crescere dentro l'Europa. Vogliamo un'Europa più empatica e vicina alle necessità e ai bisogni dei cittadini. capisco che al suo Esecutivo poco importi del Sud, dal momento che il cosiddetto contratto su cui è nato gli dedica solo sette inutili righe. Lo conferma anche il fatto che il Ministro per il Sud e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie guidano dei Ministeri senza portafoglio, quindi senza denari e alcuna possibilità di spesa o di incidere in qualche modo. Mi sorprende constatare che il sedicente Governo del cambiamento sia totalmente miope di fronte al fatto che nessun cambiamento può avere inizio se il nostro Paese è sempre più spaccato, viaggia a

meridionale, se Nord e Sud sono due Paesi diversi e il Sud sta tre volte peggio del Nord, se a Bagheria, in Provincia di Palermo, la mia città, un giovane su due non ha un lavoro e si è pure rassegnato a non trovarlo, beh, presidente Conte, forse il cambiamento di cui tanto parlate dovrebbe proprio partire da lì. lì. Presidente Conte, ci rifletta durante il suo viaggio verso Bruxelles e faccia in modo che il Governo che lei ha l'onore e l'onere di presiedere non sia, come teniamo, l'ennesima delusione per gli italiani. Signor Presidente, presidente Conte, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, non userò i pochi minuti a mia disposizione per declinare i modi di dettaglio con cui chiediamo al Governo di farsi nostro portavoce in Europa. I colleghi che mi hanno preceduto lo hanno già fatto egregiamente. Quello che vorrei consegnarle, Presidente, è un sentimento, nella convinzione che le azioni della politica da questa dimensione necessariamente si dipartono per poter

realizzando luoghi in cui nessuno presente in quest'Aula vorrebbe mai vivere, ma neanche trovarsi a passare per caso. È stato realizzato l'inferno in terra alle nostre porte ed è stato chiamato accoglienza. Sono state iniettate indiscriminatamente masse di diseredati in una società già in grande affanno, facendo esplodere disperazione e scontro sociale ed è stata chiamata umanità. Sono state abolite garanzie, estirpate sicurezze ed è stata chiamata flessibilità. È stato massacrato lo Stato sociale, chiamandolo austerità. Le parole sacre, tutte, le parole più sacre della nostra storia, della nostra centenaria cultura della convivenza, che davano un senso al nostro essere popolo, sono state abusate, svuotate, svilite. Oggi giacciono, forse per sempre o per molto, completamente fraintese. Abbiamo bisogno, quindi, di trovarne di nuove o, almeno, che non siano troppo logorate dall'uso pretestuoso e di parte. Perciò oggi mi limito, nella consapevolezza che non è per niente poca cosa, a consegnarle, signor Presidente, un bisogno che, fuori dalle parole che sono state bandiere delle parti, può forse aiutarci a parlare senza equivoci della nostra volontà di accedere semplicemente a quelle basilari forme di vita e convivenza che danno senso all'esistenza. Un bisogno che, nel falò delle parole sacre, ci convince, perché fa salva la nostra istintiva attenzione all'uomo, ma declinandola, com'è corretto in una comunità, all'interno del giusto equilibrio dei diritti e dei doveri. La civiltà, infatti, infatti, sa accogliere perché è garantita da una società funzionale, non teme l'equivoco dell'abuso. La civiltà sa soccorrere, perché sa di poter condividere il peso che ne deriva con la sua comunità. La civiltà sa garantire il patto sociale - peraltro iscritto nella Costituzione - ai suoi cittadini, sa cioè prendere ma sa anche dare quando è il cittadino ad avere bisogno dello Stato e la civiltà sa trattenere lo splendore delle sue nuove generazioni nella sua disponibilità. non abbiamo bisogno di altro, le affidiamo con fiducia questo sentimento. Le chiediamo di raccontare all'Europa che il vento è cambiato, che forze popolari fortemente connesse con la realtà, perché fortemente connesse con il tessuto vivo della Nazione, sono oggi le forze che la sostengono convintamente e che queste forze oggi non possono avallare riforme se non nella direzione di maggiore civiltà, cioè unicamente produttive di speranza, lavoro, dignità e che contribuiscano a creare nella Nazione un animo individuale e collettivo pacificato e inclusivo, non più a forza ma convintamente, perché finalmente libero da paure. Abbiamo bisogno, Presidente, di un Paese pacificato per poter anche e soprattutto guardare convintamente oltre i nostri confini. quell'Europa che abbiamo contribuito a fondare, ha in sé tutta la grandezza per comprenderlo. Grazie, buon lavoro.

n. 5, dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e n. 6, dalla senatrice Bernini e da altri senatori. I testi sono in distribuzione. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

il Presidente del Consiglio ha già esposte le linee di azione alle quali il Governo si atterrà nel corso del prossimo *summit* dei Capi di Stato e di Governo europei. Ho seguito attentamente il dibattito, ho letto le sei risoluzioni pervenutami. Prima di esprimere il parere su queste risoluzioni per conto del Governo, desidero aggiungere qualche riflessione sul quadro generale entro cui collocare i problemi contingenti. Anche se può apparire enfatico, ho la certezza che in Europa stiamo conducendo una battaglia civile, stiamo scrivendo una nuova storia. Non operiamo quindi per la cronaca, questa può esserci anche avversa, ma sarà costretta a riflettere sulle iniziative che stiamo intraprendendo per riconciliare l'architettura istituzionale dell'Unione europea con la politica che riteniamo necessaria per un'Europa più forte e più equa, un obiettivo del programma di Governo che la maggioranza ha già approvato all'atto del voto di fiducia. Dobbiamo, perciò, districarci dal contingente delle proposte in discussione nelle sedi comunitarie per integrarle con la nostra visione del futuro sulla quale il Parlamento verrà informato per raccogliere le sue valutazioni e il suo indirizzo. Sono passati oltre trent'anni dall'Atto unico europeo del 1987, che ha gettato le basi per l'attuazione di quell'Unione europea che aveva come obiettivo il raggiungimento dell'unificazione politica sognata dai Padri fondatori dell'Europa postbellica, considerata condizione indispensabile per la pace e il benessere delle popolazioni martoriate da due guerre mondiali. Fin dalla confluenza di questo atto solenne nel Trattato di Maastricht del 1992 è emerso che il clima di reciproca sfiducia fra Stati membri risentiva della pesante eredità del passato e l'accordo raggiunto fu un compromesso, tenuto insieme dalle promesse di benessere materiale (il rapporto Cecchini voluto da Delors) e non dal cemento di un'effettiva volontà di mettere in comune le sorti delle popolazioni europee aderenti agli accordi. Sulla base di previsioni prive di solide basi logiche, fu detto che l'euro avrebbe propiziato l'unione politica. Lo *slogan* usato allora fu *money first*, la moneta realizzata prima dell'indispensabile unione politica che avrebbe dovuto reggerla. Queste due debolezze della costruzione unitaria (sfiducia reciproca e assenza di unione politica), su cui il mio maestro Carlo Azeglio Ciampi insisteva con la sua definizione di zoppia, sono emerse sotto la spinta dell'incalzare degli eventi epocali che hanno interessato il pianeta dopo la caduta del muro di Berlino a cavallo di due millenni. Nondimeno, lo stretto nesso logico tra mercato e moneta unica resta valido e occorre operare perché diventi anche uno stretto nesso pratico. La ragione indica che sul piano tecnico esistono soluzioni ai difetti dell'accordo allora raggiunto. Sul piano politico, però, la loro accettazione richiede perseveranza e pazienza ma anche nessuna acquiescenza: quelle caratteristiche che gli elettori hanno già riscontrato nel nostro Governo sui problemi delle relazioni intraeuropee. Il debito pubblico italiano ha dietro un ingente patrimonio pubblico e privato: sette volte il PIL; una propensione al risparmio delle famiglie comparativamente elevata rispetto all'Europa e una solida economia con una componente di rilievo capace di affermarsi nella competizione internazionale.

Gli strumenti alternativi finora proposti per ovviare all'assenza di un *lender of last resort* che contrasti la speculazione e per dotare l'Unione europea di un assetto istituzionale che affronti le crisi strutturali non appaiono adeguati nei tempi di reazione e nella dimensione necessaria. Siamo fiduciosi che lo diventeranno e opereremo in tal senso. I dettagli di questa azione verranno resi espliciti nelle sedi parlamentari deputate. Le date degli incontri sono state fissate nel calendario dei lavori parlamentari. Per assolvere a un siffatto impegno ho già convocato per il 5 luglio, dopo il Consiglio d'Europa, il Comitato interministeriale per gli affari europei per concordare con i colleghi di Governo la linea futura da seguire e la divisione dei tanti compiti da assolvere. In conclusione, a nome del Governo esprimo parere favorevole sulla risoluzione di maggioranza, contraddistinta, nei documenti che mi sono stati consegnati, dal numero 3. Esprimiamo, inoltre, parere favorevole nei limiti della compatibilità con i programmi di governo sulla risoluzione contraddistinta dal numero 1, che porta la firma dei senatori Gasparri e altri sulla direttiva Bolkestein. Infine, premettendo premettendo che tutti i punti trattati nelle altre risoluzioni e quelli che ho sentito nel corso del dibattito saranno oggetto di seria considerazione, esprimo per essi parere contrario. Grazie.

che, avendo una certa pratica delle comunicazioni del Governo prima del Consiglio europeo, sono rimasto un po' colpito dall'irritualità. il ministro Savona abbia fatto senz'altro delle considerazioni interessanti - che, anzi, credo giusto che siano al centro del nostro dibattito - in termini logici forse la sua

penso che in quest'Aula e nel Paese non ci sia nessuno italiano che possa dire di essere contrario a questi principi di riforma. Io ho una grande paura, lo dico con sincerità: temo l'approccio che noi abbiamo seguito per arrivare a questo Consiglio europeo, a partire dal doppio binario in base al quale il Ministro dell'interno fa una parte, anche nei confronti di alleati come i francesi, e il Presidente del Consiglio

che questa strategia del doppio binario e tutto quello che è successo in queste settimane ci indeboliscano. Detto questo, se la finalità è quella che voi ponete al centro della vostra risoluzione, è difficile non essere d'accordo. Vorrei invitare però i colleghi di fare una riflessione, veramente in una totale serenità: perché mai un Paese, che non è di prima accoglienza, dovrebbe accettare una condivisione di responsabilità che in termini nazionali immediatamente lo danneggia, se si accetta una visione sovranista e intergovernativa dell'Europa? Se c'è una visione intergovernativa dell'Europa, è chiaro che ciascuno si fa gli affari suoi e ciascun Governo tutela gli interessi dei propri cittadini. Solo in base ad una visione comunitaria o addirittura federalista dell'Europa è possibile ottenere quello che il presidente Conte pone come obiettivo dei suoi dieci punti. *(Applausi dal Gruppo PD)*. anche rispetto all'opinione pubblica, ed essere coerenti nella logica perché - scusate - se accettiamo una visione in cui ciascuno è responsabile dei propri confini nazionali, in base a che cosa volete che il signor Orban si faccia carico di coloro che arrivano a Lampedusa? E infatti ho il timore che in qualche modo il signor Orban non se ne faccia affatto e temo che questo, purtroppo, lo vedremo nelle prossime ore. Sono pessimista sull'esito, però vorrei rivolgere alla Presidenza una richiesta.

vediamo se è possibile che non si venga in Parlamento solo alla vigilia del Consiglio europeo, ma si venga anche dopo, per spiegare quello che concretamente si è ottenuto.

auspichiamo che abbiate successo, perché se avete successo voi gli interessi nazionali in questo momento verranno salvaguardati. Temiamo però che le cose non siano così semplici e abbiamo molti dubbi che questa strategia sia la più efficace. Termino dicendo due cose. delle sanzioni e il no ad un meccanismo automatico di rinnovo delle sanzioni: è giusto e mi sembra sia anche in continuità con quanto altri Governi avevano proposto in Europa. La seconda difesa dei diritti dei nostri connazionali nel Regno Unito: anche questo è in totale continuità con quello che i presidenti Renzi e Gentiloni Silveri avevano proposto in Parlamento, per cui siamo d'accordo. Un *memento* finale: sento che ci occupiamo molto della politica degli altri Paesi, tante volte vogliamo andare dentro a ciò che succede negli altri Paesi e magari fare sponde a qualcuno che, in altri Paesi, gioca delle partite

i propositi di chi ritiene auspicabile una crisi del Governo tedesco, perché il giorno in cui non ci fosse più la signora Merkel, siamo sicuri che per l'Italia sarebbe sicuramente peggio di quello che è stato fino ad oggi.

ministro Savona in rappresentanza del Governo, visto che il presidente Conte si è allontanato, colleghi, gli incontri europei dei prossimi giorni sono cruciali per il destino dell'Unione europea e soprattutto per quello dell'Italia. Si discuterà infatti non solo della gestione dei flussi migratori, ma anche di sicurezza e difesa, di Brexit, di innovazione digitale, di occupazione e crescita, del bilancio comunitario su questi argomenti il Governo è stato piuttosto silente. Le ragioni della permanente campagna elettorale sono state più rilevanti del dibattito su come rimodulare le spese dell'Unione per sostenere la crescita economica e aiutare chi ha più bisogno. Avete ancora una volta usato l'arma della propaganda più becera e pericolosa, avete usato in modo spregiudicato e cinico la vita delle persone per alzare il prezzo delle trattative in Europa. Già in passato è stata usata anche da altre forze politiche questa strategia, in cambio di una maggiore flessibilità finanziaria. Si tratta di una scelta miope, che non risolve né l'uno né l'altro problema.

Chi governa ha il dovere di tenere il nostro Paese lontano da certe pulsioni, che voi invece alimentate ogni giorno. Il Governo, a cui spesso viene dettata la linea da Ministri diversi dal Presidente del Consiglio, si presenta in Europa dopo aver dato una bruttissima e imperdonabile immagine di sé. Siete riusciti, nel breve tempo di poche settimane, a inimicarvi la parte di Europa con la quale invece dovremmo dialogare, a meno che l'alternativa non sia di farlo con uomini come Orban, che non vogliono cambiare l'Europa, vogliono distruggerla. Nonostante i buoni rapporti e l'identità di vedute sovraniste con il ministro Salvini, il presidente Orban non ha accolto nemmeno un migrante di quelli previsti dalle quote. tipici conflitti tra sovranisti: i migranti non li voglio e te li tieni tu. Su questi presupposti, con il rilancio addirittura da parte dei Paesi di Visegrád del tema del respingimento dei rifugiati che provengono dai Paesi dell'Unione europea, è legittimo ritenere che quei dieci punti illustrati dal presidente Conte non siano altro che un ennesimo tentativo non troverà il doveroso accoglimento in sede europea. Noi non abbiamo dubbi: stiamo dalla parte di chi crede in un'Europa diversa, più unità e solidale, non dalla parte di chi coltiva l'incubo nazionalista. Temevamo che l'Europa si potesse disgregare per l'euro, adesso temiamo che l'Unione europea si possa sgretolare sull'immigrazione. Voi davvero pensate di poter fermare la disperazione di migliaia di persone che fuggono da guerre, povertà e violenze mostrando il pugno di ferro con i disperati in balia del mare? Voi credete che chiudere un porto non aprirà altre e più pericolose vie d'accesso al nostro continente? Voi davvero sostenete l'idea che aprire degli *hot spot* lontano dalle nostre coste, lì dove ogni basilare diritto umano è regolarmente violato, possa pulire la coscienza? Voi davvero ritenete che militarizzazione il nostro mare, da secoli crocevia di incontri di culture, ci renderà un Paese migliore, in grado anche di cambiare in meglio la Comunità europea? Noi di Liberi e Uguali crediamo fortemente di no. Noi pensiamo che questo sia il tempo del coraggio; coraggio nel difendere l'idea che nessuna cifra vale la vita di un uomo, coraggio di ricordare che a un naufrago non si chiedono i documenti, si tende la mano. Voglio cogliere questa occasione per ringraziare l'ammiraglio Pettorino, che ha corretto una vergognosa affermazione del Ministro dell'interno che istigava a commettere il reato di omissione di soccorso. Il comandante della Guardia costiera ha dichiarato: noi agli SOS rispondiamo sempre, è un dovere morale prima che giuridico. Al di là di ciò, va affermata con chiarezza la necessità di una nuova politica europea riguardante l'immigrazione, fenomeno destinato a durare nel tempo. Pensate che anni fa si calcolavano in due milioni gli africani pronti al balzo verso l'Europa; ora, secondo recenti stime, sono addirittura raddoppiati e si parla di quattro milioni. Il diritto d'asilo, sancito da trattati internazionali, richiede una legislazione comune, accordi riguardanti vie d'accesso sicure, accoglienza degli aventi diritto da parte dei singoli Stati; occorre investire maggiormente in politiche di adeguata e dignitosa accoglienza, di integrazione, di inclusione reale. Affrontare il problema solo in termini di sicurezza è miope, oltre che foriero di politiche aberranti. Serve in particolare un salto di qualità da parte dell'Unione europea nei confronti del continente africano nel suo insieme, con politiche più coerenti. Sia chiaro, l'Italia è, insieme ad altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, in una posizione insostenibile a causa del regolamento di Dublino. Siamo i primi - e colgo l'occasione per ringraziare la nostra europarlamentare Elly Schlein per lo straordinario lavoro che ha fatto a Bruxelles su questo tema - a credere che vada superato il criterio del primo approdo. Siamo i primi a chiedere a Francia, Spagna e Germania, ma anche a tutti gli altri, di mettere da parte gli egoismi e le rendite di posizione, in favore di una vera condivisione dei problemi del nostro continente. Oggi ci sarà una grande mobilitazione, promossa da più di 200 associazioni in oltre 140 piazze in Europa, per la *European solidarity*, alla quale mi sento di aderire convintamente. che giudizio si può dare del fatto che i partiti che sostengono questo Governo hanno votato contro o si sono astenuti sulla proposta del Parlamento europeo di rivedere quel regolamento, superando il criterio del primo approdo e sostituendolo con la redistribuzione dei richiedenti asilo in tutti e 27 gli Stati membri? Sui giornali, in roboanti dichiarazioni e a colpi di *tweet* di grande impatto chiedete che l'Europa cambi; ma lì dove quel cambiamento può avvenire siete clamorosamente assenti o contrari. Siete ancora una volta forti con i deboli e deboli con i forti: questa è la cifra del vostro Governo. Difendete con forza questa proposta domani al Consiglio europeo. Parlate di invasione, di emergenza, di orgoglio nazionale finalmente ristabilito; sarebbe invece il caso di parlare di spaventosa e incomprensibile retorica della paura. Basta *slogan*, basta. Migliaia di uomini, donne e bambini sono morti in questi anni al largo delle nostre coste. Forse per voi sono un po' di clandestini in meno. Per noi erano esseri umani.

noi siamo assolutamente consapevoli del fatto che da domani questo Governo ha un impegno importante, perché questo Governo e il Presidente del Consiglio rappresenteranno la nostra Nazione in un vertice europeo importante, che potrebbe essere una svolta

questo non si può fare, quello non si può fare e noi non ci rassegnavamo ad avere un ruolo di passacarte e a sottostare a ciò che decidevano, di volta in volta, la Germania o la Francia. Avevamo la certezza di aver perso una cosa a noi molto cara: la sovranità nelle decisioni di ciò di cui ha bisogno la nostra Nazione. Quindi siamo contenti che questo Governo abbia messo nell'agenda politica europea l'Italia e il problema dell'Italia, perché siamo consapevoli che, quando c'è un problema, bisogna trovare il modo per poterlo risolvere. Bene anche la scelta coraggiosa del ministro Salvini di non fare più attraccare le navi ONG, che spesso agiscono fuori da ogni norma nazionale e internazionale. Quindi il cambio di passo lo sentiamo e abbiamo anche sentito molte parole che sono musica per le nostre orecchie. Detto questo, dobbiamo entrare nel merito di ciò che questo Governo presenterà in Europa e dobbiamo dire che, sui dieci punti che l'Italia presenterà, alcuni sono da noi condivisibili, mentre altri non lo sono per niente. E, anche in quei punti che condividiamo, non ne condividiamo poi la ricetta, non ne condividiamo la soluzione. Siamo contenti che, ad esempio, ci siano gli *hot spot* sulle coste dell'Africa. Siamo anche soddisfatti che il Presidente del Consiglio abbia capito che il tema centrale non è il Trattato di Dublino; non ci sembrava dello stesso avviso quando è venuto qui a fare il suo discorso di insediamento, quindi è

quindi sappiamo che questa non può essere una soluzione, perché soltanto l'8 per cento di chi arriva in Italia ottiene lo stato di rifugiato. Il nostro problema centrale sono i clandestini e usiamo questa parola perché il linguaggio è una convenzione ed è bene che sul nostro linguaggio non arretriamo. Quindi il problema sono quei 200.000 clandestini che continuiamo a mantenere e quelle altre centinaia di migliaia che sono usciti dal circolo dell'accoglienza: persone che vivono nel nostro Paese, ma che sono bombe sociali, persone che non sappiamo cosa fanno per vivere e spesso commettono reati, spacciano, rubano, violentano. Sono persone invisibili per le leggi, ma i cittadini italiani ne sentono molto bene la presenza e ne hanno paura. Dalla paura all'ostilità, come sappiamo, il passo è molto breve. Il problema quindi non è di ottenere dall'Europa la spalmatura anche dei clandestini, clandestini, ma è altro e ci può essere soltanto una soluzione: quella del blocco navale, proposta da sempre da Fratelli d'Italia. Credo che questo Governo sia consapevole che il prosieguo della costruzione dell'Europa non sarà l'euro, ma sarà proprio la questione degli immigrati. Quindi noi diciamo al Presidente del Consiglio e a tutto il Governo che debbono abbandonare la timidezza, che debbono andare in Europa con più coraggio e che dovrebbero portare al vertice europeo il tema della protezione dei nostri confini. Devo dire - e mi dispiace che non ci sia il Presidente del Consiglio - che averlo visto ieri al tavolo col presidente francese Macron, che ha insultato l'Italia e che ha definito noi italiani «vomitevoli», mi ha lasciato e ci ha lasciati basiti. Mi permetto di dare un consiglio al Presidente del Consiglio: è bene che vada alle cene e agli aperitivi solo con chi rispetta l'Italia e gli italiani, soprattutto perché la Francia - e di questo dovremmo essere tutti consapevoli - ha grossissime responsabilità. La Francia che fa accoglienza con i porti degli altri e soprattutto con i porti italiani; la Francia che ha fatto scelte scellerate, come attaccare la Libia di Gheddafi, non certo per uno spirito umanitario ma per interessi economici e per sostituirsi all'Italia nel rapporto privilegiato che abbiamo sempre avuto con la Libia.

Quindi il tema centrale della soluzione è quello di difendere i nostri confini, come sta facendo una parte dell'Europa, come stanno facendo altri Paesi del Mediterraneo come la Spagna e la Grecia.

con un blocco navale in accordo con le autorità locali. Il Governo Prodi, in accordo col Governo albanese, fece un blocco navale per impedire la partenza dei barconi. Se ne faccia una ragione anche chi sta in quest'Aula, la sinistra che oggi critica tantissimo i blocchi navali. Consiglierei al Presidente del Consiglio, prima di partire, di fare una telefonata a Prodi, che magari, da questo punto di vista, potrebbe dare degli utili consigli. consigli. Il blocco navale si può e si deve fare, attraverso un accordo con le autorità libiche, un blocco navale concordato. Sappiamo che l'Unione europea ha tutte le argomentazioni politiche ed economiche per convincere le autorità locali, come ha già fatto con la Turchia per fermare la rotta balcanica. Quando il problema c'era, ma non disturbava l'Italia, disturbava la signora Merkel, si è risolto dando 6 miliardi di euro alla Turchia, che ha fermato la rotta balcanica. Con la stessa strategia, se mettiamo in campo risorse ingenti, come 6 miliardi in quattro con le autorità libiche, sicuramente otterremmo la loro collaborazione per istituire il blocco navale. Ricordiamoci sempre che oggi l'Italia partecipa a 114 missioni internazionali, che poco hanno a che fare con i nostri problemi, ma l'Italia c'è. Abbiamo, allora, il diritto di chiedere una missione che risolva i nostri problemi e i problemi degli italiani? Aggiungo un'altra considerazione. Noi spendiamo 5 miliardi di euro per l'accoglienza; questi soldi potrebbero essere spesi meglio, potrebbero non andare a ingrassare alcune cooperative, potrebbero non essere usati per tanti albergatori che non avevano clienti e che, con il *business* dell'accoglienza, sono tornati a fare soldi. Potremmo spendere questi soldi dandoli alla Libia, anche per non avere le coscienze sporche di sangue e per salvare coloro che partono da quelle coste, perché il Mediterraneo è troppo pieno di morti.

scorsi. In un contesto in cui tutti controllano i propri confini, controllare i confini della nostra penisola significa soltanto il blocco navale. con un dispiacere, perché nei dieci punti non abbiamo trovato una parola sui rimpatri. questo Governo se le vuole tenere? Il Governo dovrebbe cogliere lo spirito di Fratelli d'Italia, della sua opposizione patriottica. Siamo persone serie, non siamo contro tanto per essere contro; siamo a favore di tutto ciò che serve all'Italia e agli italiani e per questo ci saremo sempre. Ci vuole coraggio: andate, chiedete il blocco navale e chiedete di istituire un fondo europeo per i rimpatri. È per questo che il voto di Fratelli d'Italia sarà espresso attraverso l'astensione.

tentiamo di ricondurre a ordine la nostra discussione, che è stata importante. Dopo l'intervento della senatrice Garnero Santanchè, considerata anche la dimensione pubblica del dibattito, è bene ricordare che di qua c'è l'opposizione, che dovrebbe essere anche di là, ma non è ben chiaro. Bisognerebbe, altresì, ricordare che l'intervento del Presidente del Consiglio di oggi, importante, segue settimane di fatti che nulla hanno a che vedere con le intenzioni e gli indirizzi che oggi è venuto a esprimere. Ministro Savona, noi vorremmo mandare al prossimo Consiglio europeo un Governo forte e autorevole, per il bene del Paese; credo sinceramente che noi non ne disponiamo. Non lo dico sulla base di un pregiudizio o per parte presa rispetto alla contrapposizione politica; lo dico perché questo Governo ha profondamente equivocato sul concetto di forza e autorevolezza. Avete pensato che lasciare in mare qualche nave con un po' di disperati, evocare sporadicamente non certo la chiusura di porti, ma l'indisponibilità all'attracco (che è una cosa molto diversa) vi avrebbe portato a quel tavolo in una posizione di forza. In realtà, non c'è né forza, né autorevolezza. Ministro, con tutto il rispetto che si deve al Governo della Repubblica, mi permetta un'osservazione: avete equivocato tra il concetto di attenzione e quello di rispetto. Avete ottenuto attenzione, ma non avete ottenuto rispetto. Sono due cose profondamente diverse e la credibilità del nostro Paese in questo senso è messa a dura prova. Nessuno ha intenzione di minimizzare le difficoltà che ha di fronte questo Governo, a partire da quella degli sbarchi, ma è un errore clamoroso sovrapporre le politiche di governo dei fenomeni migratori con le politiche di governo degli sbarchi, l'uno è un fenomeno limitato e circoscritto, l'altro necessita di una strategia vera. Vorrei dire Vorrei dire al Presidente del Consiglio che non gli saranno più consentiti alcuni elementi di ambiguità anche rispetto alle posizioni che intende esprimere per conto del Paese. Oggi il presidente Conte ha fatto riferimento a una gestione europea degli sbarchi e siamo d'accordo; ha fatto riferimento a una revisione dell'accordo di Dublino e siamo d'accordo; ha fatto riferimento al processo di *relocation* e redistribuzione e siamo d'accordo; ha fatto riferimento all'intervento dell'Europa nei Paesi di partenza e siamo d'accordo. Chi glielo dice al presidente Conte

nel CARA di Borgo Mezzanone - spero che il nostro Presidente, che è di quelle terre, abbia il tempo di visitarlo - ci sono 700 profughi sorvegliati dall'esercito. Attorno a questo CARA ci sono 7.000 persone accampate senza soluzione di continuità. Oltre queste 7.000 persone, c'è il cosiddetto ghetto: 20.000 persone

l'unica dimensione del rapporto è individuare le responsabilità. Queste persone sono lì da molti anni, molto più di Gentiloni Silveri, molto più di Renzi, molto più di Letta. È importante che gli italiani sappiano che non avete intenzione di mettere mano *(PD)*. È importante che gli italiani sappiano che abbiamo intenzione di affrontare solo i problemi provocati da una settimana a questa parte. Là ci sono migliaia di persone. L'invito che vi faccio quando affrontate le politiche di gestione dell'immigrazione, non solo le navi che Toninelli e Salvini provano a fermare, perché dovreste una risposta agli italiani e dovreste una risposta, come l'abbiamo dovuta dare noi a quelle decine di migliaia di persone. Di fronte a quegli accampamenti che fate? Integrazione o ruspa? Oppure tutte e due? Oppure nessuna delle due? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Oppure continua questo teatrino, per cui si viene qua

si stanno ponendo una domanda: qual è il vero volto di questo Governo? Ministro Savona, qual è il vero volto di questo Governo? Sui temi economici, dell'occupazione e del lavoro, che porterete in Consiglio europeo, il volto è quello del ministro Tria, che invoca il rispetto dei conti pubblici e, con grande realismo, certifica l'inapplicabilità del «mitico» contratto, o è quello delle mance di Di Maio e Salvini? Lo dovete dire voi,

Qual è la visione che offre alle nuove generazioni di questo Paese? E non mi riferisco solo alla polemica di una generazione che dovrebbe campare - secondo voi - di reddito di cittadinanza. Mi riferisco al fatto che, quando, alcuni giorni fa, avete tolto dalla riforma della scuola la chiamata per competenza, avete detto a questo Paese una cosa molto precisa: fine della richiesta dei profili rispetto all'adeguatezza e alla competenza; rimane solo un criterio - sto facendo cronaca - quello

Riprendete la politica di rafforzamento del reddito di inclusione. Riprendete la politica di sostegno agli investimenti del piano Industria 4.0. Queste misure, sì, hanno prodotto risultato. Oppure possiamo continuare così: possiamo continuare senza deporre le armi di distrazione di massa, che oggi si chiamano mezz'ora di connessione Internet; ieri la scorta di Saviano; il giorno prima la lotta ai rom; il giorno prima ancora la pistola fumante sul comodino di casa. *(Applausi dal Gruppo PD).* Andiamo avanti sperando che gli italiani su questo aprano un credito, e non discutiamo - come non abbiamo fatto in quest'Assemblea fino a oggi di imprese, di lavoro, di famiglie, di sofferenza. Penso che sia un onere che sentite in carico almeno quanto noi. Ministro, concludo richiamandola se posso - alla Costituzione, sulla quale il Presidente e tutti voi avete giurato nel momento dell'incarico a questo Governo. La Costituzione vi ricorda che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, la persona prima del cittadino, la persona prima della cittadinanza, i diritti inviolabili dell'uomo. Su questo a nessuno è concesso di soprassedere. E credo che questa Assemblea dovrebbe considerare il diritto a non morire davanti alle coste del nostro Paese come diritto inviolabile dell'uomo. Su questo ci sia un'assunzione definitiva delle politiche del Governo. È tempo di chiudere,

colleghi senatori, colleghe senatrici, visto che ho poco tempo a disposizione, avendo dato spazio ai colleghi, non entro nel merito dei vari temi che saranno trattati nel Consiglio europeo, né tantomeno delle tematiche previste all'interno della risoluzione perché sono state abbondantemente discusse. Nell'esprimere un voto favorevole, ci permettiamo come Gruppo di mettere in evidenza alcune sottolineature. Di sicuro, ci troviamo di fronte a un momento storico particolare per il futuro dell'Unione europea. L'obiettivo è farci ascoltare in Europa di più di quanto sia avvenuto sinora. Solo se ci ascolteranno, se ascolteranno l'Italia, allora sì che eviteremo quella disgregazione di cui prima abbiamo sentito parlare. Siamo d'accordo con le parole del presidente Conte che, durante il dibattito sulla fiducia, ha parlato di prevenzione, e cioè dobbiamo prevenire questa disgregazione e l'Italia può giocare un un ruolo assolutamente centrale. Per noi, se si ascoltano l'Italia e il Governo italiano, allora sicuramente salviamo anche l'Europa. Non penso sia una questione solo di "prima i francesi", "prima i maltesi", "prima i tedeschi" o "prima gli italiani". È soprattutto, in Europa, "prima i popoli", poi le *élite*, le banche, la finanza e tante altre

quando dice che il vero europeista è colui che vuole cambiare i trattati dell'Unione europea, colui che vuole cambiare l'Europa. Su questo noi siamo assolutamente d'accordo e vogliamo che l'azione di Governo vada in questa direzione. E finora il Governo si è mosso bene. Tutti parlano, e noi sentiamo discutere di propaganda. No! Abbiamo visto il Governo in azione. Si è mosso bene, senza sudditanza politica e psicologica, senza timore nei confronti dei nostri *partner* europei, mettendo al centro dell'azione gli interessi dei cittadini italiani. E non è un caso che l'Italia partecipi finalmente a un vertice in una posizione di forza, da protagonista. Altro che isolamento! Non diamo retta alle sirene della minoranza. Viviamo nel mondo al contrario: più ci attaccano, più vuol dire che abbiamo ragione e dobbiamo andare avanti. E infatti ci chiamano tutti, da tutto il mondo: ambasciatori, statisti, da tutte le parti. quindi significa che l'Italia è ritornata, sì, al centro dell'attenzione. Ci stiamo ritagliando un ruolo diplomatico di mediatori tra le varie posizioni che ci sono in Europa. Questo è quello che la minoranza non ha ancora capito o che finge di non capire. per dare maggiore equilibrio all'interno dell'Europa stessa, addirittura anche oltre confine, vista la nostra posizione anche con gli Stati Uniti e di dialogo tra Stati Uniti e la Russia stessa, quindi l'Italia che ritorna finalmente protagonista.

al Consiglio europeo, attenzione a non accettare contentini di alcun genere, perché siamo sicuri e certi che Germania e Francia *in primis* tenteranno ancora una volta di imporre il loro modello di *governance* su tutta l'Europa. Noi dobbiamo mantenere la barra dritta e portare l'Europa sulla strada del buonsenso,

onorevoli colleghi, mi dispiace pronunciare la dichiarazione di voto a nome del Gruppo Forza Italia in assenza del presidente Conte. Farò come se ci fosse, certa che il ministro Savona saprà ben rappresentare la nostra posizione. Il Consiglio europeo giunge in un momento delicato della vita comunitaria. Come sappiamo, i

Quindi, presidente Conte, non pensi a scambi al ribasso. Nessuno pensi di cedere in cambio di qualche pacca sulla spalla - ad esempio sull'unione bancaria - dando così il via alle proposte franco-tedesche che sono penalizzanti per i nostri istituti di credito, o magari per qualche margine irrisorio sulla spesa per realizzare qualche misura assistenziale e/o elettorale, come il reddito di cittadinanza. Come il ministro Savona sa perfettamente, i mercati non lo perdonerebbero. Quello che quindi appare - e che purtroppo non è diverso dalla realtà dei fatti - è come il Governo arrivi in confusione a questo appuntamento e come l'agenda italiana - ammesso ne esista una - rischia di essere solo

La profonda diversità tra le anime di questo Governo - un ircocervo, a voler essere buoni - e le dichiarazioni disarmoniche dei suoi membri e dei membri della maggioranza che lo sostengono sono la dimostrazione di come si navighi alla giornata. Non c'è un'azione propria dell'Esecutivo, ma tutto è piuttosto affidato all'iniziativa dei singoli Ministri, alle loro sensibilità e alle loro più o meno nobili esigenze. È questo un limite assoluto, che non dà credibilità a lei, signor Presidente del Consiglio, né all'Esecutivo che presiede, né tantomeno al nostro Paese. Questa babele di linguaggi e questo procedere in maniera difforme sono quindi un problema e un grave danno che si riverberano negativamente su tante, troppe questioni. Vale per il capitolo del bilancio comunitario, vale per la necessità, non più rinviabile, della riforma dell'Unione europea e dell'eurozona e vale anche - e soprattutto - sulla questione migranti. Anche su questo, presidente Conte, il suo Governo suo Governo è totalmente schizofrenico. Macron insulta l'Italia e gli italiani e lei tiene incontri riservati nell'elegante cornice della Casina Valadier, mentre il Ministro dell'interno ricambia tono su tono gli apprezzamenti. Se non si tratta di parti in commedia, evidentemente qualcosa non torna. Mi chiedo però con quale credibilità ci si presenta oggi a parlare nei consessi europei di immigrazione quando nel contratto di Governo e nelle sue dichiarazioni programmatiche non ci sono una riga o un'idea del futuro sul Mediterraneo, su come affrontare le sfide e le problematiche epocali che ci provengono da quell'area del mondo. I dieci punti famigerati - mi consenta - sono tutto tranne che una visione del domani e in questo scenario europeo, con questi equilibri e con la sua debolezza, rischiano di essere un libro dei sogni. Le emergenze - gestione dei flussi in testa - vanno certamente affrontati. Il problema andava posto nelle sedi comunitarie e di questo dobbiamo dare atto al Ministro dell'interno. non è sufficiente sapere che in Europa hanno finalmente compreso che non possiamo restare soli - semmai lo hanno compreso - o che la Sicilia e l'Italia non dovranno mai più essere i soli *hotspot* del Mediterraneo.

lo *spread* sia ben alto. Lei ha di fatto rivendicato come un successo la conclusione del vertice informale sui migranti che si è svolto domenica a Bruxelles, ma ciò corrisponde a una verità parziale, per non dire a una bugia. Infatti, se è vero che tutti i *leader* seduti al tavolo concordano, almeno ufficialmente, almeno a parole, sul fatto che i flussi devono essere gestiti a livello comunitario, è altrettanto vero che non c'è un minimo accordo su come farlo. Nelle bozze che filtrano e nelle sue dichiarazioni, si parla genericamente di spezzare il modello di *business* dei trafficanti - cosa sacrosanta - dell'ipotesi di centri di smistamento di migranti fuori dall'Unione europea

Lo stesso vale per la Libia, sui cui destini sarebbe interessante sapere cosa pensa il suo Governo. Tra i Paesi extra UE disponibili ce ne sono alcuni - guarda caso - sulla rotta balcanica. Il perché forse lo potrebbe chiedere alla cancelliera Merkel, la quale ha di sicuro ben presente quali sono le priorità del suo Paese: si parla, infatti, dell'Albania e della neodenominata Repubblica macedone del Nord, interessate a entrare nell'Unione europea e ancor più ad avere un po' di risorse. Trionfalismo e dichiarazioni a parte, è è chiaro che non c'è un minimo di intesa e di disponibilità, al netto del Marocco, dei Paesi riviersachi della sponda Sud. Ma passiamo al capitolo risorse.

Numeri alla mano, è del tutto evidente che l'impegno di spesa vero riguarda il corridoio balcanico e non l'area che più direttamente interessa l'Italia. Non si è chiesto perché? Forse anche questa spiegazione potrebbe chiedere alla Germania o all'Austria. Per inverso, da quanto emerge non c'è una sola posta economica prevista per il corridoio libico, nonostante le aperture del commissario al Bilancio Günther Oettinger e gli appelli del presidente Tajani. Allo stato, ci sono solo buone intenzioni. Eppure, per affrontare l'emergenza che arriva dal Mediterraneo e che più ci interessa e ci tocca da vicino, servono circa sei miliardi di euro. Chiudere la cosiddetta rotta libica significa intervenire soprattutto in Paesi come il Ciad e il Niger, i cui tassi di crescita demografica sono impressionanti e fanno il paio con la fame e la miseria. Quanto alla riforma di Dublino non si faccia illusioni: è in alto mare e non sarà facile che si trovi una conclusione nel breve periodo. Illustre Presidente, non potrà quindi bastare, e non potrà essere considerato in alcun modo un successo per l'Italia e per il suo Governo,

Italia lo invochiamo a gran voce. Crediamo che sia giunto il momento che l'Italia impegni con serietà i Paesi europei, nel loro interesse, allo sviluppo concreto di un piano per i Paesi da cui originano i fenomeni migratori. È questo anche il senso profondo della risoluzione che il nostro Gruppo ha inteso presentare ed è la ragione per cui non possiamo votare a favore di risoluzioni che non rappresentano la realtà delle cose,

in queste ore ci troviamo a vivere un momento storico difficilissimo per il futuro del nostro Paese e dell'intera Europa. Per la prima volta, però, dopo tanti anni, abbiamo finalmente un Governo che ha dimostrato che con autorevolezza

Ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi e non posso non sottolineare come si sia parlato di marchette. Ed è assurdo parlare di marchette per un Governo che oggi inizia a fare i suoi primi provvedimenti. Ma da assurdo diventa surreale se a parlare di marchette è il Partito Democratico! Per favore, colleghi, terminiamo questa seduta in maniera dignitosa. Siamo di fronte a un bivio, a due scenari completamente alternativi su temi fondamentali quali l'immigrazione, la sicurezza comune e la lotta alla povertà, che dipendono dall'esito del Consiglio europeo di domani e dopodomani.

l'obsoleto e iniquo principio dello Stato di primo ingresso; un'Europa che consideri il Mediterraneo come frontiera europea di comune responsabilità e lavori in Africa con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni per creare centri internazionali di protezione e assistenza ai richiedenti asilo e canali legali e sicuri di accesso all'Europa. Solo in questo modo sarà possibile stroncare sul nascere la disumana tratta degli esseri umani e porre fine ai terribili viaggi della speranza e all'ecatombe dei barconi della morte. L'alternativa alla strategia europea per l'immigrazione proposta dal Governo italiano è lasciare tutto com'è. Avremo quindi un'Europa sempre più divisa e litigiosa, che chiuderà a cascata le frontiere nazionali da Nord a Sud e inizierà a sgretolarsi pericolosamente, continuando a scaricare il fardello della gestione dei migranti sui Paesi rivieraschi di primo approdo, a partire dall'Italia. Chi arriva in Italia, a Malta o in Grecia arriva in Europa. al tema della difesa, una nuova politica europea dell'immigrazione deve significare - come si è detto - anche un controllo congiunto e condiviso della comune frontiera marittima mediterranea. Questo deve essere il primo obiettivo concreto di una nuova politica comune di sicurezza e difesa. Gli altri obiettivi devono essere quelli di intensificare la lotta ai trafficanti di esseri umani e incrementare il necessario lavoro di *intelligence* condivisa antiterrorismo, sia nel dominio reale che in quello virtuale; potenziare gli strumenti di contrasto alle crescenti minacce informatiche e, pur mantenendosi saldamente nel solco dell'Alleanza nordatlantica, riavviare la preziosa cooperazione con la Federazione russa in materia di pace, sicurezza e lotta al terrorismo. Importantissima, infine, è l'implementazione di una cooperazione europea in campo di armamenti, perché consentirà di eliminare molti sprechi nelle spese per la difesa. Con i risparmi di questi sprechi, poi, e con l'organizzazione europea della difesa potremmo fare quegli interventi che sono fondamentali per la lotta alla povertà. Una razionalizzazione della spesa consentirebbe di disporre di più soldi da investire in un'altra difesa, quella della dignità, del lavoro, della salute dei cittadini italiani ed europei. Resta dunque più che evidente l'assoluta urgenza di difendere il popolo italiano dalla minaccia della povertà, di dichiarare guerra alla povertà e all'esclusione sociale, intraprendendo coraggiose politiche di sostegno al reddito, a partire dall'attuazione della nostra proposta di reddito di cittadinanza, che esiste in tutti o quasi i Paesi europei. politiche finanziabili anche con la razionalizzazione della spesa per la difesa. Ritengo quindi che l'impegno del Governo sui temi del Consiglio europeo in materia di immigrazione, sicurezza comune e lotta alla povertà risponda agli interessi del popolo italiano e quindi dell'Europa tutta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

Senatore Marcucci, la ringrazio perché sarei stata io a dire al senatore Romeo che questa indicazione sarebbe venuta da parte della Presidenza e del rappresentante del Governo. Si stava chiedendo al senatore Gasparri se, in virtù di quanto il Governo è pronto a chiedere, in base alla risoluzione, sull'integrazione da fare, è d'accordo.

e sono d'accordo con quanto ha detto il Governo. Io l'ho presentata al Governo e quindi accetto l'integrazione all'intero testo chiesta dal ministro Savona e insisto per la votazione. Mi pare questa la procedura che si segue in Senato.

Faccio fatica a essere preciso se non c'è un po' di silenzio. delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi,

e il disegno di legge n. 473, recante misure urgenti per il potenziamento e l'estensione del diritto d'inclusione e per favorire l'occupabilità dei suoi beneficiari, hanno il numero di firme previste per essere fatti propri dal Gruppo,

Presidente, signori Ministri, onorevoli senatori, non posso esimermi dal trasmettervi l'emozione toccante che ho esperito sabato mattina, nella mia terra, il Friuli-Venezia Giulia, durante la cerimonia di resa degli onori solenni e tumulazione di 100 caduti in terra di Russia. A Cargnacco, in provincia di Udine, riposano uomini (direi piuttosto ragazzi) che partirono per assolvere il proprio dovere in nome della Patria e che per la Patria morirono. È un luogo dove una lapide in bronzo ricorda coloro che erano stati mandati tra i ghiacci della Russia con le scarpe di cartone. Sabato mattina a Cargnacco hanno fatto ritorno 100 salme di soldati morti nelle steppe, 100 urne avvolte nel Tricolore, portate in braccio da 100 militari in armi.

Sono state deposte nel piazzale del sacrario per la cerimonia religiosa, per essere poi trasportate con l'ultimo abbraccio dei commilitoni nel tempio sacro. La ritirata di Russia è finita qui, nella grande cripta della Madonna del conforto nel sacrario di Cargnacco, in Friuli-Venezia Giulia. Dei 100 caduti, solamente sei avevano un nome che ha permesso di rintracciare le famiglie per la restituzione delle spoglie; famiglie di anziani

del dovere, di appartenenza e in nome di tali valori ha immolato il tesoro più prezioso, la propria vita. Come non commuoversi? Come non ricordarli con il dovuto onore? La ricerca e il rimpatrio dei caduti sono stati realizzati dal commissariato generale per le onoranze ai caduti del Ministero della difesa, in collaborazione con l'ambasciata

si tratta di aree in cui si combatté la famosa seconda battaglia difensiva del Don, ove transitarono le nostre truppe della 8a Armata. Il generale Alessandro Veltri, commissario generale per le onoranze ai caduti, ha dichiarato che l'attività del commissariato generale nel campo della ricerca e del recupero dei caduti è incessante e continuerà sempre con lo stesso spirito. Su un totale di più di 90.000 caduti accertati e dispersi nei territori dell'ex Unione Sovietica, solamente 11.840 hanno fatto ritorno in Italia grazie al commissariato generale; altri 80.000 corpi sono

e di Nazione, cadendo a difesa dei propri valori indossando una divisa. Informo che sul portale del Ministero della difesa il Commissariato generale per le onoranze ai caduti ha creato un *link* dove i familiari possono richiedere informazioni dei loro cari dispersi nelle terre dell'Est. Grazie per l'attenzione.

Signor Presidente, oggi ricorre il trentottesimo anniversario della strage di Ustica. Trentotto anni di attesa per una verità che sembra non arrivare mai e a cui manca ancora un tassello fondamentale:

al risarcimento dei parenti delle vittime non bastano. Cercare la verità è doveroso per rendere giustizia alle 81 vittime, ai loro familiari e al Paese intero. Per questo è fondamentale, e lo è stata, l'attività dei magistrati, per continuare a indagare su una tragedia che troppe volte si è cercato di camuffare con tesi improbabili e insostenibili. Apprendiamo da fonti di stampa la notizia per cui i magistrati della procura della Repubblica di Roma interrogheranno un ex membro dell'equipaggio della USS Saratoga, che la sera del 27 giugno 1980 era in servizio sul ponte della portaerei americana e la cui testimonianza potrebbe forse aprire uno spiraglio sulle effettive responsabilità di quella notte. Al di là di questo, mi auguro che ci possano essere ulteriori passi significativi verso la verità. Noi non smetteremo di ricordare quella notte e di coltivare la memoria di questo Paese, per quelle vittime, per i loro parenti e per noi stessi, perché esercitare la memoria vuol dire non dimenticare il passato, cercare la verità

anche da parte nostra c'è un ricordo, che vuole essere particolare in quest'Aula, della strage di Ustica, di cui ricorre proprio quest'oggi trentottesimo anniversario. Guardando l'orologio che è dinanzi a me, ricordo che trent'anni fa, tra otto minuti, alle ore 20,08, 81 persone si stavano per imbarcare su quel volo, tra cui 11 bambini e 4 membri dell'equipaggio. Quando si trovarono, alle ore 20,59, sul cielo di Ustica, nel braccio di mare tra Ponza e Ustica, i radar di Roma ne persero le tracce e quell'aereo cadde in mare con il suo carico di morte. anni di distanza noi non sappiamo ancora qual è la verità; noi non sappiamo esattamente che cosa è avvenuto. Io credo che sia importante - mi rivolgo ai membri del nuovo Governo, pensando e ritenendo

in particolare per desecretare gli atti che sono ancora coperti da quella coltre di nebbia che non è ancora stata spazzata via. E allora, se ricerchiamo la verità, la dobbiamo cercare tutta; e per farlo dobbiamo compiere questo passo, per rendere veramente onore a quelle persone, non in un momento semplicemente suggestivo d'Aula, ma per andare incontro a loro, ai loro familiari e soprattutto a quella verità che l'Italia stessa chiede. Ed è una verità a cui anelano anche le nostre coscienze. Abbiamo chiesto tante volte, più volte, anche magari a Governi esteri, di fare chiarezza su tanti episodi, e a giusta ragione lo abbiamo fatto. Noi vorremmo Noi vorremmo mettere la parola «fine» a questa lunga notte della Repubblica. A buona ragione abbiamo chiesto quindi questa questa verità. Spero e mi auguro che lo si possa fare. Lo dobbiamo alle vittime, lo dobbiamo ai loro familiari, lo dobbiamo alle nostre coscienze, lo dobbiamo all'Italia. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, membri del Governo, il 29 giugno 2009 a Viareggio un incidente ferroviario ha causato la morte di 32 persone: uomini, donne e bambini portati via dal fuoco mentre si pensavano in sicurezza nelle loro case. Signor Presidente, sono trentadue anime che chiedono piena giustizia. La sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale di Lucca ha già individuato dei colpevoli: tra questi, Mauro Moretti, allora amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Moretti che liquidò la strage di Viareggio come uno «spiacevolissimo episodio», affermazione che ricorda quel «destino cinico e baro» in riferimento a un'altra tragedia toscana, quella del Moby Prince. Moretti che poi fu addirittura proclamato da Giorgio Napolitano nientemeno che cavaliere del lavoro, uno schiaffo per le vittime e i familiari di una strage che si poteva e si doveva evitare si fosse investito in sicurezza. Noi insistiamo che a Mauro Moretti venga subito revocato il cavalierato. Ciò che è successo in questi nove anni è rappresentativo del peggio della cialtroneria *made in Italy*: i tentativi di scaricare le responsabilità, la latitanza dello Stato, il depistare la verità, il tutelare i poteri forti invece che le vittime, la codardia e la mancanza di dignità nell'assumersi la responsabilità e di chiedere scusa dinanzi a tanta sofferenza. Presidente, la sofferenza e la sete di giustizia non vanno in prescrizione e noi riformeremo questo istituto. Manifestiamo la nostra vicinanza a tutti i familiari delle vittime, all'associazione «Il mondo che vorrei», il cui presidente, Marco Piacentini, ha perso moglie e due bimbi piccoli. Manifestiamo altresì la nostra vicinanza al ferroviere Riccardo Antonini, che è stato licenziato da Ferrovie dello Stato, reo di aver prestato gratuitamente la propria consulenza all'Associazione familiari delle vittime. Questa è una vergogna. *(Applausi dal Colleghe e colleghi, il vagone che è deragliato il 29 giugno 2009 è simbolo di quel sistema economico neoliberista che ha come unico obiettivo il profitto e non il benessere dell'uomo. Non dimentichiamo Viareggio, non dimentichiamo la nostra umanità.

e sul quale cronache recenti stanno evidenziando i suoi appelli all'ascolto. Quello di cui siamo convinti è che ogni cittadino deve, in ogni ambito, sentirsi sicuro, sorretto e seguito dallo Stato. Anche in questo senso il Ministro si è espresso chiaramente: «Ho ascoltato il video del carabiniere Casamassima su Facebook e sono disponibile a parlare con lui». «Quanto al trasferimento» dice ancora il Ministro «può essere stato deciso anche soltanto per tutelarlo. Questo dobbiamo approfondirlo». È in questo senso e in questo contesto che, insieme ai colleghi del MoVimento 5 Stelle e della Commissione difesa, intendiamo procedere. Chiederemo a Riccardo Casamassima di informarci sulle sue vicissitudini, al fine di raccogliere dettagli utili alla ricostruzione di una vicenda che va sicuramente chiarita e approfondita, in un'audizione conoscitiva e informale, per ascoltare e capire prima di emettere qualsiasi giudizio.

Mi riferisco a 48 milioni di euro di soldi pubblici che sarebbero dovuti essere sui conti di un primario partito del Governo, la Lega, e che su questi conti non sono stati trovati. Sono soldi frutto - secondo una sentenza di primo grado - di una truffa commessa ai danni dello Stato. Questa interrogazione è stata presentata al Ministro della giustizia il 17 aprile; nelle more della formazione di nuovo Governo (non c'era il nuovo Governo) abbiamo atteso, ma ora basta. C'è il nuovo Governo, c'è il Ministro della giustizia: è tempo di fare chiarezza e di rispondere ai quesiti posti La seconda interrogazione, a mia prima firma, la è stata presentata ai Ministri della giustizia e dell'interno e riguarda fatti che sono oggetto di un'inchiesta del settimanale «L'Espresso», pubblicata il 7 giugno 2018, e si riferiscono, in particolare, ai flussi finanziari nei confronti di una ONLUS, «Più Voci», che è presieduta dal tesoriere della Lega. Sono fatti meritevoli di attenzione e su questi chiediamo, con le interrogazioni che ho richiamato, se il Governo ne sia a conoscenza, quali valutazioni ne dia e quali azioni il Governo e i Ministri interrogati intendano adottare, su circostanze - lo ripeto - che sono allarmanti, inquietanti e assolutamente rilevanti, perché riguardano un tema molto delicato e sensibile, come il finanziamento della politica. Sono doppiamente rilevanti per altri due motivi: il primo è che riguardano un primario partito di Governo e il suo rapporto di correttezza nei confronti dello Stato e delle normative di finanziamento della politica; il secondo motivo è che il capo politico di questo partito è il Ministro dell'interno; gli rivolgiamo, insieme al Ministro della giustizia, alcune domande e il ministro Salvini ha il dovere di rispondere e di fare chiarezza. Per tramite suo, signor Presidente, rinnoviamo al Governo l'invito a rispondere rapidamente a queste interrogazioni e le chiediamo di farsi parte attiva in questo senso, sulla base di una profonda convinzione: che rispondere a un atto di di sindacato ispettivo è un atto di rispetto doveroso, non solo nei confronti di questo Parlamento, ma innanzitutto nei confronti dei cittadini.